un lutto che colpisce tutti, perché Andrea Purgatori è stato uno dei più bravi giornalisti italiani. A lui si devono tante inchieste su teatri di guerra, teatri di guerra, tante inchieste sui fenomeni del terrorismo, della criminalità organizzata e su grandi fatti di cronaca. Se diciamo «il muro di gomma» lo si deve a lui, perché indagò sull'aereo abbattuto sopra il cielo di Ustica dopo alcuni anni e scoprì, con il giornalismo d'inchiesta, la verità su quel muro di gomma che era stato costruito attorno a quella tragedia.

irrobustire la libera informazione e il giornalismo di inchiesta. Per questo ho ritenuto, signora Presidente, di dire queste parole, perché penso davvero che sia una di quelle notizie dolorose, ma assolutamente da condividere anche in consessi come questo.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, devo ammettere che non capisco proprio gli argomenti che portano il Governo italiano a volersi intestare il triste vanto di essere il primo al mondo a vietare preventivamente i prodotti a base di carne coltivata, prodotti che stiamo ancora studiando, per i quali si stanno raccogliendo dati scientifici, a cui stanno contribuendo i ricercatori delle nostre università (l'Università di Trento, Tor Vergata, l'Università di Napoli, l'Università di Torino). A pensarci è un corto circuito pazzesco, perché qui si tratta di vietare le applicazioni di quello che stiamo ancora studiando. Ma, se stiamo studiando, significa che non sappiamo; non sappiamo l'impatto, non sappiamo la percezione del pubblico, le ricadute, la qualità. Se non so, come faccio a decidere che non li voglio? Qual è la qualità legislativa di una simile decisione? Se il fastidio è nel chiamare questi prodotti "carne", mi associo a quanto detto ieri dal senatore Spagnolli: trattandosi di alimenti che sembrano analoghi, sotto il profilo nutrizionale, alla carne da macellazione, possiamo chiamarli in altro modo, se questa è la condizione per non proibirli. Oggi con voi vorrei trattare di sei elementi contradditori relativi a questo primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata. Il primo elemento riguarda la sorprendente esclusione degli studiosi dalle audizioni su una materia che ha forti componenti scientifiche e tecnologiche. Vedete, sono in Senato da dieci anni e continuo a credere che studiare sia l'elemento indispensabile per capire la realtà e le sue evoluzioni e per prendere decisioni individuali e collettive che riguardano la vita di tutti noi. Già ieri la collega Aurora Floridia ha denunciato come le Commissioni 9a e nell'esaminare il disegno di legge, abbiano limitato le audizioni in presenza, escludendo incredibilmente gli studiosi e i ricercatori del Paese attivi in questo ambito, ai quali è stato chiesto di inviare delle memorie scritte, quando sarebbe stato utile ascoltarli, sentirli, frequentarli e capire cosa vedono in quella direzione, sulla quale stanno spendendo la loro vita. Per nulla? Per niente? Avranno delle motivazioni. Perché non ascoltarli? Fanno parte del nostro Paese e delle nostre università. Tra l'altro, pensate che proprio gli studiosi italiani gli studiosi italiani non auditi sono quelli che hanno scritto un mese fa su «Nature Biotechnology» un articolo che ha proposto alla comunità scientifica mondiale di contribuire a costruire sulla carne coltivata un consenso scientifico volto a evitare eventuali, anche se del tutto improbabili, fughe in avanti, che possano porre problemi di ordine sanitario o bioetico. Quindi ci si interroga insieme. La senatrice Floridia ha ricordato ieri come l'aggettivo "sintetico" sia del tutto inappropriato per descrivere i prodotti di cui stiamo discutendo oggi. Quindi il termine va emendato e davvero spero che tutti noi staremo attenti a non riproporre questa trappola linguistica. Come secondo punto vorrei analizzare con voi la motivazione per la quale il principio di precauzione, invocato a fondamento della legge in discussione, sia aberrante rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento europeo del 2002.

che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole. Se ci sono motivi validi o potenziali rischi, la messa in atto di procedure precauzionali può essere di grande aiuto sociale. Ma attenzione, il principio di precauzione non può essere usato o sbandierato come una clava, come uno strumento retorico per sollevare paure irrazionali o guidate da gruppi di interesse. proposito cito per tutti la memoria agli atti delle Commissioni inviata dall'Associazione nazionale dei biotecnologi: i prodotti per i quali si intravede un rischio che possa prefigurare l'attivazione del principio di precauzione in Europa oggi non esistono

rischi che possono essere indagati e gestiti in fase autorizzativa sui *novel food*. L'altro aspetto che la memoria dell'Associazione nazionale dei biotecnologi ricorda ricorda è che i divieti in via di introduzione non rispettano i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato all'invocazione del principio di precauzione, che non può diventare un principio di limitazione. Anche ieri, sempre su questo, vari senatori hanno sottolineato come la legge sia inutile oggi, perché vieta qualcosa che è già vietato, e sarà inutile domani,

europea ne autorizzerà il commercio all'interno dell'Unione e, una volta autorizzati, sappiamo bene che non potranno essere fermati alla frontiera. L'esito dell'inserimento del principio di precauzione è che con questa legge e con questo principio le nostre imprese non potranno produrre una serie di elementi, non potranno cimentarsi, non potranno innovare. Non è vero che non si blocca la ricerca, perché si sta dicendo ai ricercatori Il terzo punto riguarda le le narrazioni terroristiche sui bioreattori e sulle staminali pericolose. Il senatore Spagnolli ieri, a proposito delle narrazioni sulla carne coltivata che si produce in bioreattori, ha ricordato che anche yogurt, birra e vino, anche a livello casalingo, si producono in bioreattori. Aggiungo che, grazie ai bioreattori, oggi abbiamo l'insulina, ma anche i vaccini e gli anticorpi monoclonali che ogni giorno salvano migliaia di vite. Sempre il senatore Spagnolli ieri ricordava che per spaventare i cittadini si sono dipinte le biotecnologie a base di cellule staminali come pericolose. Attenzione, qui si entra proprio nel mio campo di lavoro:

e molto altro). Perché dovremmo dunque averne paura, quando sarà uno scienziato di Trento o di Roma ad usarle per fare una crocchetta di pollo come quella dei *fast food* che il nostro corpo digerisce in poche ore?

che riporta un aumentato rischio cardiovascolare in seguito al consumo di alimenti processati e ultralavorati, ma - attenzione! - ci si rifà a prodotti da carne da macellazione,

secondo lo IARC, quella più pericolosa e sicuramente cancerogena. Tuttavia, nessuno immagina di vietarli, perché - ed è giusto ricordarlo sempre ai cittadini - è la dose che fa il veleno, quindi la frequenza e la quantità del consumo. In ultimo, il quinto punto che mi porta a discutere con voi è la discriminazione che il disegno di legge opera tra aragoste e bovini: per le prime la carne coltivata è consentita, per i secondi è vietata. Il divieto per la carne coltivata vale solo per gli animali vertebrati, ma possiamo produrre carne da echinodermi, ricci di mare, cefalopodi e molluschi. Forse i rischi paventati per carne coltivata

la pasta con i ricci di mare coltivata può avere la grazia di essere considerata *made in Italy*, o forse i pescatori diretti di cozze, calamari, polpi, aragoste e ricci non godono presso il Governo di sufficiente ascolto? O magari sono semplicemente più attrezzati a guardare al futuro e all'innovazione come fattore di sviluppo. Credo che il Governo debba fornire le ragioni tecniche alla base di questa differenziazione. Infine, ultimo punto, vi è la libertà di scegliere come nutrirsi. Questo disegno di legge, a mio avviso, si configura come un ennesimo arretramento scientifico, economico e culturale del nostro Paese, che mortifica i nostri ricercatori, tarpa le ali ai nostri imprenditori più innovativi, limita la libertà di scelta dei cittadini che vorrebbero poter provare, se certificati come sicuri, questo tipo di prodotti. Non sono pochi questi cittadini: ho sentito ieri nella discussione ripetere che "solo" il 18 per cento dei cittadini italiani vorrebbe consumare prodotti a base di carne coltivata. Ebbene, stiamo parlando di 10 milioni di italiani a cui questa maggioranza sta per limitare ideologicamente la libertà di scelta alimentare. Trovo sia offensivo e paternalistico considerare i cittadini come eterni bambini in svezzamento, rispetto ai quali lo Stato si arroga il diritto di decidere cosa possano assaggiare e cosa no, in nome di un richiamo improprio ad un principio di precauzione applicato in maniera tombale, quando invece per sua natura è temporaneo e rivedibile. In conclusione, il mio e il nostro dovere nelle istituzioni è difendere i cittadini da chi li ritiene incapaci di comprendere i benefici della ricerca, difendere gli studiosi da chi ne disconosce il lavoro e l'eccellenza, difendere gli imprenditori da chi vuole limitare la loro libertà di impresa, cioè quella di svolgere nelle loro aziende e con i loro soldi le attività che ritengono, quando queste non nuocciono ai cittadini. Da studiosa e da senatrice, sento anche il dovere di manifestare la mia ferma opposizione a una deriva culturale pilotata da portatori di interesse del mondo agroalimentare, che vogliono impedire a nuovi attori economici di affacciarsi sul loro stesso mercato, facendo dell'Italia il campione mondiale del terrore della conoscenza. Questa è una responsabilità che graverà su questa istituzione parlamentare e su quanti tra noi, a sprezzo di ogni ragionevolezza - mi sia consentito - anche del ridicolo, sceglieranno di assecondare con il proprio voto una narrazione avulsa dalla realtà. Signor Presidente, invece noi della Lega ringraziamo il Governo per essere intervenuti tempestivamente sull'ultima trovata *green* della finanza mondiale, ossia questa carne sintetica, che adesso, per renderla più digeribile all'opinione pubblica nazionale e mondiale, chiamano "carne coltivata". Già la parola "*green*" più la sento e più mi fa venire l'orticaria, quindi va bene un intervento da parte del Governo, perché posso capire che ci siano alcune *lobby* internazionali che naturalmente intendono fare affari con la transizione energetica e con la scusa del cambiamento climatico. Non è che mi stupisce o ci stupiscono queste cose. Sappiamo che il mondo è mosso prevalentemente da interessi economici, dal cosiddetto dio denaro, quindi di cosa ci dobbiamo stupire? Lo sappiamo. Come non ci dobbiamo neanche stupire che queste multinazionali sostanzialmente finanzino delle azioni volte a spingere gli Stati nazionali a investire su queste nuove tematiche. Non è una novità e l'abbiamo detto più volte che anche i cosiddetti ecoteppisti che vanno a parlare dell'ambiente non sono certo giovanotti veramente animati da questo spirito ambientalista. Anche perché poi abbiamo scoperto - e l'abbiamo letto sui giornali che appartengono ad una rete internazionale *(Applausi)* finanziata da un fondo californiano con sede a Beverly Hills, creato da un ex collaboratore di Bill Gates. Quindi complimenti all'anima ambientalista di questi giovanotti.

(sostanzialmente un governo mondiale non eletto), ha dichiarato che, mentre l'umanità si dirige ulteriormente verso un futuro *post* carbonio, il popolo deve accettare che il mangiare carne e la proprietà privata sono cose semplicemente insostenibili. Ecco, il fatto che questo Governo non si faccia dettare l'agenda politica da questi signori *(Applausi)* è un fatto politico rilevante. Grazie al cielo, c'è un Governo di centrodestra. premesso - ed è sacrosanto, lo dico - l'insegnamento che va fatto a tutti, a partire dai ragazzi, ossia che bisogna rispettare l'ambiente, che esso va tutelato, che bisogna diversificare le fonti energetiche, investire nelle fonti rinnovabili, rispettare la natura prendendosi cura del proprio territorio, cercando di ridurre i consumi e i materiali più inquinanti: è tutto sacrosanto, giusto e ho detto più volte che sono contento che nelle scuole si insegni questo. Però, vedete, non e addirittura credere che il cambiamento climatico sia un fenomeno del tutto nuovo e che sia tutta responsabilità dell'uomo, come se l'irradiazione solare, i cicli planetari sono sostanzialmente i cicli astronomici legati alle variazioni solari), il peso delle orbite non abbiano alcuna influenza. A proposito di scienza - visto che si parla molto di scienza in quest'Aula - sembra che il periodo caldo romano, quello medievale, la piccola glaciazione, il processo di ritirata dei ghiacciai, non siano mai esistiti. Ecco il clima della Terra è sempre cambiato e ce lo dice il senatore a vita Carlo Rubbia, fisico italiano e vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984, senatore a vita dal 2013, per il quale chiedo un applauso forte *(Applausi)*, perché dobbiamo anche ricordarci di chi ha studiato, è in quest'Aula e dovrebbe insegnare a tutti. Si vuol far credere addirittura che fra poco non ci sarà più il cibo disponibile, che saremo costretti a vivere in zone desertificate a causa del riscaldamento globale. Tra l'altro, l'Europa causa dell'8 per cento delle emissioni di CO₂ nel mondo, mentre tutti gli altri continenti sostanzialmente se ne disinteressano. A proposito, a me hanno sempre insegnato che la CO₂ è alla base della vita, non è un inquinante e, anzi, ha effetti positivi per le foreste tanto decantate e per l'agricoltura. credere che se in Europa compreremo solo auto elettriche, se andremo tutti a 30 chilometri orari, se metteremo i pannelli fotovoltaici ovunque e se rinunceremo soprattutto a mangiare la carne, perché gli allevamenti bovini inquinano, e mangeremo invece un bel panino con la carne sintetica o con gli insetti, salveremo il Pianeta. Perdonatemi, ma è semplicemente contro ragione e contro ogni logica; questo sì che è semplicemente ridicolo. Ma non mi preoccupano certi discorsi fatti in quest'Aula, poiché la politica la conosciamo bene da tantissimo tempo. Quello che mi preoccupa invece è che questa nuova religione - perché di religione si tratta e non di scienza - venga venga insegnata nelle nostre scuole ai nostri ragazzi. Che vada avanti il Governo, perché questo non è solo un aspetto di un provvedimento, ma un aspetto culturale che va assolutamente contrastato. *(Applausi)*. Complimenti al Governo, ai relatori e a tutta la maggioranza per il coraggio che abbiamo avuto di di denunciare questa ennesima vergogna *green*.

gode indubbiamente di un fascino particolare. Forse, lo aggiungo per l'ennesima volta, si poteva e si doveva affrontare questo argomento in un altro modo. non lo dico perché mossa dalla certezza che quanto stiamo discutendo abbia delle evidenze scientifiche comprovate e incontrovertibili, ma perché, se nel corso della nostra storia avessimo affrontato l'innovazione tecnologica e scientifica così come oggi la state affrontando, l'Italia sarebbe arrivata sempre seconda a qualsiasi altro Paese. C'è da dire, per amore di verità, che il populismo ci ha fatto arrivare secondi più e più volte, proprio su argomenti e questioni simili a quella che stiamo affrontando oggi. Lo ha fatto quando si è trattato di discutere di OGM, della commercializzazione della cosiddetta cosiddetta farina di insetti, quando si è dovuto affrontare il tema della *xylella*. In tutti questi casi, la totale assenza di serietà e di attenzione verso la ricerca, ma aggiungerei anche l'utilizzo di questi temi in termini propagandistici, ha generato un dibattito il più delle volte non all'altezza della situazione, animato dalla contrapposizione ideologica, che non dovrebbe appartenere alle istituzioni che ci onoriamo di rappresentare, ma che dovrebbe portarci a fare lo sforzo di non fermarci all'apparenza, bensì di esaminare in profondità la natura delle cose. colleghi, quando è stato incardinato il provvedimento in esame, ho letto con attenzione, come sempre mi capita di fare, la relazione illustrativa che precede l'articolato. Devo confessarvi che in quella relazione ho trovato tutte le ragioni per le quali questo provvedimento, a mio avviso, risulta essere totalmente privo di senso. Cito testualmente: «Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti». «In alcuni Paesi extraeuropei sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti. Negli Usa, la Food and drug administration ha dato l'ok alla cosiddetta carne sintetica, alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio, cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo». Approfitto per ricordare all'Assemblea e a chi ci segue da casa che non esiste alcun prodotto sintetico, quando si parla di questa materia. Almeno su questo aspetto la maggioranza ci ha ascoltati e ha accolto l'emendamento che modifica sia il testo che il titolo ed ha corretto, infatti, in tutto l'articolato, il termine «carne sintetica» con il termine corretto, che è «carne coltivata» o o «a base di colture cellulari». Sempre nella relazione viene specificato che «va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carte coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale sia ancora oggetto di ricerca» scientifica. Al netto delle posizioni che ognuno di noi può avere, rispetto alle ricerche e al lavoro di analisi su questa tipologia di prodotti alimentari, a me pare però chiara una cosa: stiamo parlando di prodotti su cui la scienza e la ricerca stanno effettuando studi, indagini e analisi. Lo scrivete chiaramente, come ho ricordato, lo mettete nero su bianco, prima di citare una sfilza di studi contrari a questa pratica. Forse è per giustificare il senso di questo provvedimento. Quanto stiamo discutendo è oggetto di una ricerca che si sta compiendo a livello internazionale e che indubbiamente avrà una proiezione futura che vedrà coinvolta, com'è giustamente scritto nella relazione, prima ancora che l'Italia, l'Unione europea.

e quello di rischio sono analoghi ai prodotti già autorizzati. In pratica, se questi prodotti dovessero essere autorizzati dall'EFSA, questa discussione sarebbe del tutto inutile, come qualsiasi discussione riguardante l'approvazione e la commercializzazione di un farmaco,

Non voglio entrare nel merito della questione, cosa che farò a breve. Voglio capire le ragioni che spingono un Governo a formulare un provvedimento di questo genere. Vedete, se ci fosse stato un pericolo concreto all'orizzonte, forse vi avremmo anche seguiti. Ma noi siamo di fronte ad una situazione nella quale la ricerca sta andando avanti, nella quale gli eventuali progressi sarebbero in capo ad enti e istituzioni sovraordinate e sovranazionali, nella quale l'Europa già vieta ciò che voi volete vietare con questo provvedimento e nella quale, nel caso in cui l'Europa dovesse autorizzare questi prodotti, il divieto previsto dal dal provvedimento andrebbe in frantumi perché in contrasto con i trattati europei. Ecco, di fronte a tali premesse io vi chiedo: perché questo provvedimento? Credo che la risposta, in realtà, sia molto semplice. Voi avete la necessità di agitare e fissare, per l'ennesima volta, una bandierina. Io quasi preferirei che raccontaste che ci diceste chiaramente che, dopo aver rinominato il Ministero dell'agricoltura Ministero della sovranità alimentare, avevate il bisogno di continuare ad alimentare uno *storytelling* che piace ad un mondo affine al vostro, che vi permetta di riempire le pagine dei giornali e di nascondere che, da mesi a questa parte, non abbiamo mezza risposta concreta ai veri problemi che gli italiani stanno vivendo in questi mesi! E nessuna risposta state dando agli allevatori, con questo provvedimento. Ma su questo dirà meglio, dopo di me, il collega Franceschelli. Io dico chiaramente che è un gran peccato, perché in quest'Aula potevamo discutere seriamente delle eventuali opportunità o degli eventuali pericoli derivanti da una pratica come quella della carne coltivata. Lo avremmo fatto dialogando, innanzitutto, con allevatori e coltivatori, con la comunità scientifica, con chi quotidianamente lavora in questo ambito. Lo avremmo fatto provando a spiegar loro la complessità di questa materia, provando a costruire insieme una strategia che non danneggiasse la nostra economia, ma che quanto meno permettesse all'Italia di non isolarsi. Proprio questo, infatti, è il pericolo più grande: con questo provvedimento si otterrà solo di fermare gli investimenti e la ricerca nel nostro Paese. Quale investitore, infatti, sceglierebbe l'Italia per fare ricerca, a fronte delle sanzioni previste in questo provvedimento? Il risultato sarà molto semplice e lo abbiamo già visto in passato. Faranno ricerca al confine, negli Stati europei dove Governi seri non sentono il bisogno di vietare ciò che è già vietato o di normare ciò che non si conosce. Il risultato sarà scontato: mentre tutto il mondo potrà elaborare dati e fare ricerca, noi diciamo un secco no ideologico. E lo facciamo il nome della difesa del *made in Italy*. Mi sento di dire che, forse, è esattamente il contrario, perché noi distruggiamo completamente la possibilità di far nascere un'imprenditoria

comprendere, approfondire e imparare e lo dico avendo stima e rispetto delle preoccupazioni di intere filiere, di amministratori locali e dei colleghi di maggioranza e opposizione, relative ai risvolti che la questione potrebbe avere. Tuttavia, se dovessi usare una frase che sintetizza il mio pensiero, prenderei senz'altro in prestito quella usata dalla senatrice Cattaneo in occasione di un interessantissimo convegno organizzato proprio qui in Senato: «Studiare è meglio che vietare» *(Applausi),*e lo sottolineo. Non devo certo ricordare quanto lustro abbia dato e continui a dare al mondo della ricerca la senatrice a vita Cattaneo in rappresentanza del nostro Paese, ma direi che dentro il titolo di quel convegno possa essere sintetizzato bene quello che forse sarebbe il caso di fare prima di lanciarsi in fantasiose iniziative: studiare, capire e agire. *(Applausi)*.

a punto questo provvedimento abbiamo ascoltato i due milioni di cittadini che hanno firmato la petizione di Coldiretti contro i cibi sintetici; abbiamo ascoltato i 3.200 Comuni italiani che hanno approvato gli ordini del giorno contro carne e alimenti sintetici; abbiamo ascoltato le Regioni non solo quelle governate dal centrodestra - che hanno approvato iniziative legislative contro il cibo sintetico, anche quella Regione in cui fino a poco tempo fa faceva l'assessore l'attuale *leader* del Partito Democratico, che ha votato in favore di un ordine del giorno contro il cibo sintetico. *(Applausi)*. Come funziona? Quando è il centrodestra che promuove questa iniziativa, non si può fare; quando invece si è liberi di ascoltare le voci dei territori, ovviamente li si ascolta. Vediamoli, allora, tutti i motivi che ci portano a dire che questo provvedimento va approvato e va nella direzione giusta. Abbiamo già sentito parlare delle certezze sulla salute. Ebbene, non abbiamo certezze che gli alimenti sintetici siano salutari, anzi, tra le tante fonti che anche la senatrice a vita Cattaneo e altri colleghi citavano, ci siamo dimenticati però di citare la FAO

che attenzione particolare merita l'uso di componenti biologici come fattori di crescita e ormoni da origine animale o non animale, in quanto queste molecole biologicamente attive potrebbero interferire con il metabolismo e sono state associate allo sviluppo di alcuni tumori.

Per condurre ad un'adeguata valutazione dei rischi per gli alimenti a base di cellule è essenziale raccogliere una quantità sufficiente di dati e di informazioni scientifiche necessari per la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio». Ribadisco che non è il Governo a dircelo, l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO. È giusto quindi rifarsi a uno dei principi europei fondamentali, che è quello della precauzione, per cui in assenza di evidenze scientifiche è giusto fermarsi,

più di me - che i contadini sono i *designer* del panorama, perché dove non ci sono non c'è panorama e non c'è territorio che cresce bene. Dove diminuisce il lavoro nei campi si perde qualità e specificità. Un altro elemento da sottolineare è la qualità. Per noi la bellezza del mondo sta nella diversità e non nella standardizzazione e nell'omologazione. La cerchiamo, questa diversità, nei nostri cibi, l'andiamo a cercare in ogni Regione, in ogni territorio e in Italia vengono milioni di turisti a cercare questo. Immaginiamoci quante persone verranno a cercare *hamburger* e bistecche tutte uguali, con lo stesso sapore dal Giappone alla Spagna. La nostra carne è frutto di quello che mangiano i nostri animali, rispetto a dove pascolano, rispetto a quello che respirano e a dove vivono, rispetto alle 7.000 specie vegetali che in Italia, e solo in Italia, nascono e crescono. In quale laboratorio volete trovare tutta questa ricchezza? Dove volete trovare questa specificità? Tutto questo, infatti, è figlio della nostra unica biodiversità. È grazie a questa diversità che l'accesso all'alimentazione in Italia è aperto a tutti, perché qualunque cittadino in Italia si può rivolgere ad un produttore che conosce, di cui apprezza la qualità, dove può andare a cercare e trovare anche un risparmio economico, però mangiando bene. In questo non siamo gli Stati Uniti, dove pochi mangiano bene ed altri, soprattutto i più poveri, sono costretti ad attingere a cibi assolutamente non di qualità, con terribili conseguenze sulla salute: le percentuali sull'obesità americana non ve le devo certo raccontare io. E ancora, l'Italia si basa sulla filiera di produzione: c'è chi coltiva, chi alleva e pesca, c'è chi trasforma, magari in più processi, e c'è chi distribuisce. Ognuno ha e gestisce una parte del valore che questo processo determina. Il laboratorio garantisce solo il grande produttore, chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato. Noi in Italia rischiamo di scardinare un processo sociale tipicamente italiano, che parte dalla terra e arriva alla tavola, da chi coltiva a chi compra. Chi produce su larga scala e rifornisce direttamente il mercato non ha di queste preoccupazioni.

perché non è possibile ricattare nessuno sulla base del cibo e delle forniture alimentari. Nessuno può essere escluso dal mangiare, nessuno può essere ricattato per fame. Questa non è una visione fantasiosa: guardate quello che sta succedendo col grano proprio in questi giorni e in queste ore in Ucraina, dove la Russia, negando l'accesso ad alcune vie di rifornimento, tiene o cerca di tenere alcuni Paesi legati a sé sulla base di un ricatto alimentare. Siamo proprio sicuri di voler regalare questi poteri - o, almeno, questa possibilità - a laboratori (a quali laboratori, peraltro?) di qualche contadino, di qualche impresa agricola oppure delle grandi multinazionali

che possa svolgere il suo ruolo senza influenze delle multinazionali e che possa liberamente indagare sicuramente sulla validità degli alimenti sintetici, ma anche capire i giusti tempi e le loro criticità. che la ricerca possa concentrarsi, direi anche e soprattutto, per aiutare i Paesi in via di sviluppo, mettendoli nelle condizioni di avere una loro autonomia agricola e alimentare. intervento da dove l'ho cominciato e mi rivolgo ai colleghi forse ancora incerti, in particolare tra i banchi dell'opposizione. Ascoltate non Marco Scurria, ma le organizzazioni degli agricoltori, ascoltate i territori, ascoltate i cittadini, ascoltate soprattutto il buon senso, perché sarebbe retorico citare gli oltre 5.000 prodotti tipici italiani che amiamo, regaliamo, assaggiamo e valutiamo e di cui siamo orgogliosi quando andiamo all'estero, perché sappiamo che sono rappresentativi della nostra identità culturale e nazionale.

non abbiamo proprio bisogno di laboratori che sfornano carni, alimenti e mangimi senza sapore e forse anche senza senso. La collega prima diceva che rischiamo di arrivare secondi; invece con questo provvedimento l'Italia e la nostra Nazione arrivano primi, perché mettono un paletto sulla corretta alimentazione e sulla corretta ricerca scientifica. Se Feuerbach ci ricordava che siamo quello che mangiamo, io, noi, non vogliamo essere uomini sintetici.

Signora Presidente, i diversi punti di vista che sono emersi sono tutti degni di nota, ma, contrariamente a chi sostiene che è meglio studiare anziché vietare, noi siamo dell'idea che sia meglio studiare molto approfonditamente e circostanziatamente prima di autorizzare. Difatti, siamo dell'idea che gli scienziati e la scienza in generale restino la più straordinaria opportunità di sviluppo della vita, a partire dalla salute. È proprio per questo che dobbiamo proteggerli dal compiere frettolosi passi in avanti contribuendo con azioni e cautele concrete ad evitare di commettere errori. È una prospettiva in cui, in un Paese come il nostro, nel quale c'è una certa diffidenza per l'innovazione artificiale in campo alimentare, sapere che il legislatore ha privilegiato precauzionalmente la tutela della salute contribuisce a sensibilizzare e a promuovere sani stili di vita. Perciò portiamo convintamente in approvazione, stante la sua adeguatezza, il testo in esame, auspicando che vi sia una condivisione più ampia della maggioranza di Governo.

Mi sono riservato soltanto la replica, anche perché la collega Cantù era stata particolarmente esaustiva nella relazione e nella presentazione del documento. Ho Ho ascoltato tutti gli interventi, soprattutto quelli dell'opposizione, per cercare di capire se il nostro era veramente un provvedimento così

Credo che, anche volendo fare l'avvocato del diavolo di me stesso o del provvedimento del Governo, le motivazioni addotte in tanti interventi non abbiano fatto altro che rafforzare in me la convinzione che questo provvedimento non solo è giusto e non solo è doveroso,

che la politica deve avere una visione che guardi ai prossimi vent'anni e non al contingente? Spesso, sempre. E quante volte ci siamo sentiti dire che la politica - lo dico da sindaco - deve ascoltare i territori, altrimenti non serve a nulla? Allora, delle due l'una: o abbiamo sempre detto una serie di corbellerie e oggi quindi dovremmo smentirle, oppure ci sono entrambe le cose. C'è una visione - che può piacere o no a tutta l'opposizione

guarda caso la stessa cosa che vorrebbe fare quello che questo provvedimento contrasta. Noi siamo cittadini consapevoli. questo provvedimento trattiamo i cittadini come bambini che hanno bisogno di essere educati. Dall'altra parte, però, ci spiegano come educare quei bambini, dando una visione sola, quella del *politically correct*.

Governatori si sono espressi immediatamente a favore del provvedimento: Giani, Bonaccini, De Luca o Emiliano.

Usano una terminologia arcana? Sono irragionevoli? Pongono le loro Regioni in posizione isolazionistica? Si danno la zappa sui piedi?

Questa è una differenza di coerenza. Ho sentito parlare di cortocircuito. Non è questo forse un cortocircuito? Quando state sui territori, dite che hanno ragione gli agricoltori e quelli che, come gli agricoltori, non vogliono recidere un elemento fondamentale, che in questa Nazione si amplifica, ossia il legame inscindibile che c'è tra la terra e il piatto.

Vogliamo veramente arrivare a qualcosa di costruito in laboratorio in qualsiasi parte del mondo? Nessuno degli attuali benpensanti fautori o sostenitori di qualche *lobby* di scienziati può pensare che quello che poi è il frutto della ricerca potrà venire messo a terra nella nostra Nazione, dove i costi di produzione sono più alti e il costo del lavoro non è sicuramente competitivo, anche se ci abbiamo lavorato, rispetto ad altre Nazioni. Quei cibi verranno prodotti dove costa meno, dove non c'è alcun legame con il territorio e dove non c'è forse neanche alcun controllo.

se noi siamo quelli contro la ricerca, perché abbiamo dovuto aspettare che arrivasse Fratelli d'Italia al Governo per adottare due provvedimenti importanti come il *carbon farming*, cioè la capacità riconosciuta alle piante di trattenere la CO2, e, meglio ancora, il provvedimento sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA)? Se voi non eravate così oscurantisti, perché la stragrande maggioranza del Parlamento nella scorsa legislatura non è riuscita a farlo, nonostante ci fosse un ministro del MoVimento 5 Stelle che era favorevole alle tecniche di evoluzione assistita? Perché? Forse l'oscurantismo alberga in qualcuno di voi. Siete voi gli oscurantisti *(Applausi)*, siete voi che alla ricerca non credete e la adattate solo ai vostri fini personali o di chi vi sostiene, non certo noi. L'abbiamo dimostrato in sei mesi di governo: provvedimenti adottati subito. Non siamo forse noi quelli che dall'opposizione hanno pungolato i Governi, tutti quelli della precedente legislatura, per dire che il nutri-score, anche se era sottoscritto e firmato da oltre 300 scienziati o pseudotali, era una baggianata pazzesca e non aveva alcuna evidenza scientifica? *(Applausi)*. Non siamo stati forse noi a portare in Aula quel provvedimento, anche grazie alla lungimiranza dell'allora ministro Patuanelli, che lo fece votare all'unanimità da tutto il Parlamento? Siamo oscurantisti noi? Lì, a quei 300 scienziati abbiamo risposto che dicevano una sonora baggianata: abbiamo avuto il coraggio di dirglielo, come Parlamento. Oggi invece sembra che, se qualche scienziato è contrario alla carne coltivata, sintetica o come la chiamate, noi diventiamo automaticamente oscurantisti. No, non lo siamo, mi dispiace, lo abbiamo stradimostrato. Pertanto non mi resta altro che augurarmi che non solo la maggioranza che, anche nei suoi interventi, ha addotto questo tipo di motivazioni per votare il provvedimento ma anche, in fondo, le menti illuminate di questa opposizione possano capire che qui non è in discussione soltanto la salute pubblica. Guardate che il principio di precauzione significa avere cautela avere cautela e, visto che dobbiamo studiare prima e che studiare è meglio che vietare, ebbene, anche leggere è meglio che non farlo: non c'è un passaggio di questo provvedimento, infatti, che vieta la ricerca. Sarebbe bastato leggere il provvedimento, probabilmente. Io mi illudo che l'abbiate fatto, ma se l'avete fatto e non avete scorto che non c'è un passaggio contro la ricerca, forse avete letto male o forse qualcuno vi ha suggerito male le posizioni da tenere. Buon lavoro a tutti.

ringrazio tutti i colleghi, senatori e senatrici, che sono intervenuti in questo dibattito. Mi scuso per non essere stato presente ieri

Abbiamo espresso la posizione dell'Italia, che è quella di garantire una sostenibilità ambientale tendenziale che non sacrifichi, com'è successo in questi ultimi trent'anni, le nostre marinerie. Quindi le persone libere, quelle a cui faceva riferimento, anche del mondo della pesca, non solo vengono attenzionate dal nostro Governo, ma cerchiamo di capire a livello nazionale e internazionale come riuscire a coniugare i loro interessi

che i primi ambientalisti del nostro territorio siano proprio agricoltori, pescatori e allevatori *(Applausi)*, perché traggono banalmente la loro possibilità di vivere da quello che qualcuno pensa che nel tempo abbiano voluto distruggere o inquinare. Non mi riferisco ovviamente a qualcuno tra i presenti, perché so che questo consesso è autorevole da tanti punti di vista, certamente politico e istituzionale per definizione, ma anche per capacità di comprendere fino in fondo tutte le argomentazioni. È per questo che si dibatte e si approfondisce, credo in termini non ideologici, collega, esattamente il contrario. È stato già ricordato come questa legge sia frutto di un meccanismo che in democrazia credo sia estremamente virtuoso, quello di sussidiarietà: si parte dal popolo, si passa per le istituzioni del territorio, si arriva in Parlamento e si cerca di comporre un indirizzo che sia omogeneo alla volontà dei cittadini. Noi siamo rappresentanti dei cittadini e potremmo normare anche privandoci di quel sostegno che la Costituzione assegna, per altre funzioni, alle amministrazioni locali e alle Regioni, ma abbiamo scelto di non farlo: abbiamo scelto invece di agire esattamente in linea con quanto esplicitamente chiesto dalle istituzioni più prossime al cittadino. La sussidiarietà è una bella cosa mi chiedo, quando distinguiamo il "noi" e il "voi", se facciamo riferimento a un posizionamento che esula dalla connotazione che ci vede sedere in banchi assegnati ai partiti. Mi stupisce infatti

su carta intestata del Partito Democratico, che vede anche la firma di Fratelli d'Italia (ma dopo gli esponenti del Partito Democratico, tutti). Ebbene, è stato votato all'unanimità e chiede di vietare

i poteri forti dai quali alcuni si lasciano condizionare. Non credo però che il Partito Democratico toscano sia condizionato da Coldiretti, seppur richiamata esplicitamente nel testo, così come viene richiamata nel testo della Regione Campania e nel testo della Regione Emilia Romagna. Graziano Delrio, che ha presieduto una delle componenti più importanti del nostro quadro istituzionale, l'Associazione nazionale Comuni, sa quanto siano preparati i nostri amministratori locali, i nostri sindaci. Non credo che siano stati superficiali quando, in più di 3.000 Comuni e in maniera trasversale, hanno fatto le medesime richieste. Credo che siano degni di rispetto e non vadano definiti oscurantisti, ignoranti e nemici della ricerca. Lo ricordava il collega De Carlo poc'anzi e l'hanno fatto già altri colleghi: non c'è una sola virgola in questo disegno che inviti non a fare ricerca; anzi, la ricerca per noi è un elemento cardine del dibattito e ci mette in condizione oggi di muovere con chiarezza, per quello che ci riguarda,

L'Italia è una Nazione libera sulla ricerca: dobbiamo mantenere questa consapevolezza e invertire quella fascinazione verso Nazioni in cui la ricerca è affidata al privato. Il privato fa il suo mestiere, a volte nell'interesse dei cittadini, altre volte nell'interesse esclusivamente delle azioni della multinazionale che rappresenta. Credo che purtroppo questo sia il caso di molti che finanziano alcune ricerche al fine di condizionare il mercato e di indirizzare lo sviluppo, per esempio nel campo alimentare, di settori che avvantaggiano alcuni e depotenziano altri. Non è un caso che negli Stati Uniti ci sia un modello differente dal nostro rispetto, ad esempio, all'alimentazione. Si faceva riferimento al regolamento europeo che ci permette oggi di normare in quest'Aula. Ringrazio il collega Schillaci, autorevolissimo scienziato (su questo credo ci siano pochi dubbi), medico, rettore dell'università di Tor Vergata, preside della facoltà di medicina, autorevolissimo rappresentante della comunità scientifica, che ha fatto appello esattamente a quel principio di precauzione previsto nel regolamento, che indica nella European Food safety authority (EFSA) il soggetto che può o non può autorizzare il *novel* *food.* È lo stesso regolamento

ci siano rischi. Il diritto di precauzione ci permette dunque di normare e di dire che, finché non siamo certi che una cosa sia salubre per i cittadini italiani, preferiamo che non venga commercializzata e importata in questa Nazione *(Applausi)*, il che non vieta la ricerca, in nessun modo.

che hanno voluto dare un segnale. Tra quelle firme ce ne sono alcune di autorevolissimi rappresentanti italiani ed europei di molti dei partiti qui presenti, non solo del Partito Democratico. Ad esempio, in Regione Calabria è passata la mozione all'unanimità, con il voto di tutti, compresi il MoVimento 5 Stelle e altre forze politiche rappresentative, con cui si chiede esplicitamente

che, quando lo facevano, speravano che non ci fosse un Governo a raccogliere la loro istanza. Li voglio ringraziare e dir loro che abbiamo fatto esattamente quello che ci hanno chiesto *(Applausi)*: lo vogliamo ribadire e rivendicare con orgoglio, per varie ragioni.

sulla vicenda dell'alimentazione aprirò un capitolo a parte, perché credo che il cibo non sia solo carburante e che ci sia confusione su questo. Non mi convinco che il cibo sia solo carburante e non mi convinco nemmeno che gli esseri umani siano solo consumatori. *(Applausi)*. Siamo anche consumatori e siamo anche Prima di essere questo, però, siamo esseri umani, cittadini e persone che, a differenza di un oggetto che consuma, hanno una soggettività di scelta, data dalla capacità di discernimento unica, propria degli esseri umani, così preponderante sugli altri elementi che compongono la sfera del pianeta. Nel momento in cui guardiamo qualcosa, anche il cibo, siamo capaci di decidere e dobbiamo farlo sulla base di alcuni elementi. A mio avviso, l'elemento prioritario resta quello qualitativo, che oggi è discutibilmente applicabile a un sistema di produzione come quello finora messo in campo sulle produzioni di carni coltivate, o sintetiche,

nel senso che questa è una produzione molto rispettosa degli animali. Lei, professoressa, credo conosca i protocolli di produzione e sa che sulla vicenda delle produzioni di carne sintetica i vari passaggi prevedono pratiche particolarmente invasive, se non violente, nei confronti degli animali, comprese l'estrazione di liquido fetale

nell'ambito del Ministero della salute: vi è il rischio derivante da alcune patologie riscontrabili solo in animali

come qualcuno dice, nell'ottica del pieno rispetto della vita di ogni essere vivente, che noi invece abbiamo, ma che delineiamo e decliniamo nell'ambito di una della convivenza, che l'uomo ha visto con gli altri esseri viventi del pianeta, anche in termini alimentari, con una serenità che non credo possa essere messa in dubbio da

Noi vogliamo dare, attraverso questa norma, anche un indirizzo di natura politica: questo è vero. Per noi l'agricoltura, l'allevamento e la pesca sono elementi centrali. Noi non abbiamo normato sulla pesca semplicemente perché, al momento debba presentazione del disegno di legge, non era ancora noto che ci fosse un'evoluzione così accelerata della produzione di pesci sintetici:

luoghi, un'autorizzazione legata all'assunzione di responsabilità sugli effetti futuri che questo cibo possa produrre su chi lo assume. È una precauzione che di solito nei ristoranti italiani non viene

e che tolgono a noi risorse importanti, come imprese, e tolgono benessere ai cittadini che consumano cibi prodotti in Italia. Sempre parlando di dati empirici, qualcuno mi ha contestato un'affermazione. Io stimo tantissimo gli Stati Uniti. Ci hanno aiutato a riconquistare la libertà. Ci proteggono a livello internazionale. Almeno finché, nella ridefinizione della NATO, l'Europa non riuscirà ad avere un ruolo più incisivo, sono loro i protagonisti delle vicende internazionali. Gli Stati Uniti, però, una cosa non possono insegnarci: a mangiare.

non solo la longevità (che, per fortuna, ci vede tra i popoli che vivono di più sul pianeta e questo forse con l'alimentazione qualcosa c'entra), ma anche un dato inquietante, che vede, negli Stati Uniti,

Siamo una Nazione molto fortunata, dove la qualità è stata trasmessa grazie sicuramente alla comunità scientifica, ma, ancora prima, dalle mamme e dalle nonne, che tante volte, da ragazzini, ci spiegavano cosa faceva bene e cosa faceva male, sulla base di un'esperienza centenaria. In altre Nazioni questo non è accaduto, perché sono state condizionate da logiche di mercato e da una comunicazione molto forte. Ho letto l'allarmante ricerca di un'università statunitense che spiega come sui bambini delle classi meno agiate negli Stati Uniti influisca talmente tanto l'elemento del condizionamento alimentare che i massimi livelli di obesità si riscontrano proprio in quella fascia. Noi, invece, abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso le persone meno abbienti si trovano a mangiare meglio delle persone più ricche, perché acquistano, per ragioni di prezzo, dal produttore o dal trasformatore trasformatore e quello corrisponde alla qualità. Questo non avviene nelle altre Nazioni come gli Stati Uniti, dove invece chi è molto ricco o ricco mangia bene e chi è povero o molto povero si trova ad avere del cibo che

in termini di sicurezza alimentare, avendo noi una popolazione in crescita esponenziale, ci dobbiamo preoccupare di come riuscire a risolvere il problema dell'alimentazione del pianeta. Questo è un elemento forte che vede l'Italia protagonista perché ha una sua posizione, che ha rivendicato nel G7 e che sarà oggetto della Presidenza del prossimo anno del G7 in questo settore, che ha sostenuto alla FAO e che ribadirà in quella sede. Noi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza alimentare, con la convinzione, però, che non basta

anche mondiale divisa in due, tra i ricchi che continueranno a mangiare bene e a mangiare sano, e i poveri ai quali dare prodotti ipertrasformati, massivi e standardizzati. Non lo accettiamo culturalmente né economicamente.

c'è la possibilità di incentivare le produzioni in termini quantitativi e qualitativi. Orientiamo lì, per quello che ci riguarda, il massimo dell'impegno della ricerca; mettiamo a disposizione le nostre tecnologie, le nostre imprese. Ringrazio il presidente Meloni che si sta ponendo, verso quei Paesi, con questo tipo di approccio. E ringrazio le numerose imprese che si sono messe a disposizione per aiutare a far crescere quel Continente, cercando di risolvere a monte un problema che spesso ci troviamo ad affrontare a valle, aiutando e lavorando con l'Africa. Non ci arrendiamo infatti all'idea, che qualcuno per troppo tempo ha propagandato, che gli africani debbano lavorare per noi: noi vogliamo lavorare con loro per crescere insieme e la potenzialità sul cibo da questo punto di vista è un elemento centrale. *(Applausi)*. È stata contestata anche la sovranità alimentare come concetto. Ma la sovranità alimentare consiste nel continuare a decidere come si vuole produrre e quello che si vuole mangiare: una scelta che viene messa in discussione sempre più da aggressioni che tentano di condizionare le persone che acquistano e consumano. Questo Parlamento all'unanimità ha contrastato il nutri-score, un'etichettatura che per ragioni oggettive è esclusivamente finalizzata al condizionamento e non all'informazione. L'Italia non ha paura della ricerca, non ha paura della trasparenza: quando le persone conoscono, anche attraverso l'etichetta, che cosa mangiano, come viene prodotto, come viene trasformato, come lo si riesce a presentare,

e l'olio d'oliva tra i prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Certo, il quantitativo eccessivo di un prodotto alimentare può essere potenzialmente dannoso per la salute, ma lo è anche l'acqua

sue scelte l'Italia è tutt'altro che isolata: sul piano internazionale, in ogni contesto nel quale ci presentiamo - le dimostrazioni di questi giorni esulano dal mio e non le citerò, ma sono davanti agli occhi di tutti - su questi temi siamo protagonisti in Europa in un sistema di alleanze che divide i Paesi che vogliono cibo di qualità da quelli invece che immaginano che il cibo sia solo carburante *(Applausi),* dove, quindi, l'unico interesse è standardizzare, facilitare la produzione, distruggere le filiere produttive virtuose che abbiamo e che disegnano un equilibrio del valore ripartito tra tanti, accentrando le risorse e magari spostando le produzioni ove è più facile.

perché non si capirebbe mai che quello è cibo. Non servono gli occhi, l'olfatto o il tatto: lo si può capire solo dalla grande scritta «*This is food*». È la prima cosa che si vede nel supermercato: una grande «A» del nutri-score che ne designa la qualità;

dell'umanità, che passa per il buon cibo e non invece per i condizionamenti di chi immagina di fare *business* sullo sfruttamento delle fasce più povere della popolazione.

quando ha richiamato il documento che è stato sottoscritto dalle Regioni, dai sindaci, eccetera. Quel documento, quel manifesto di Coldiretti l'ho firmato anche signor Ministro, e l'ho firmato convintamente, perché in esso c'era scritto esattamente quello che noi abbiamo scritto nell'emendamento 1.10, che è stato bocciato

che, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare, dovrebbero essere riconosciuti «la giusta remunerazione degli agricoltori e allevatori, lo sviluppo progressivo dell'agroecologia, in particolare nelle aree interne del Paese, l'incentivazione e la valorizzazione degli allevamenti estensivi, anche al fine di ridurre il quantitativo delle importazioni di alimenti e mangimi per gli allevamenti di provenienza estera e premiare il consumo di foraggio di provenienza nazionale, di migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale, nonché l'innalzamento della qualità e della varietà dei prodotti commercializzati, a partire dalla

Ho ascoltato anche le sue parole in merito alla questione della valorizzazione della ricerca e le ho molto apprezzate. Io peraltro non ho mai usato nel mio intervento la parola "oscurantismo", mai. Ho semplicemente detto che la ricerca deve andare avanti, perché è una risorsa importante di questo Paese. Infatti, abbiamo presentato un emendamento che propone di inserire nel testo che è necessario garantire «la continuità delle attività di ricerca scientifica e tecnologica su alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e competenze».

L'ha ammesso oggi anche lei, signor Ministro, per cui basta approvare questo emendamento e lei sarà conseguente con le parole che ha appena pronunciato. E noi lo apprezzeremmo moltissimo.

isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati e il mantenimento nel nostro Paese di ricercatori e

Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi della maggioranza apprezzandone determinati aspetti. In particolare, mi riconosco assolutamente nell'italianità e nell'apprezzamento delle nostre tradizioni, specialmente di quelle alimentari e culinarie. L'ordine del giorno G2.107 in realtà va proprio nella direzione di tentare di ripristinare le nostre tradizioni originarie. Tutti ricorderete che nei vari cascinali si ammazzava il maiale all'inizio dell'inverno per poter avere sostentamento, la domenica si ammazzava la gallina e l'apporto alimentare proteico di derivazione animale era rarefatto, nel senso che era un alimento prezioso di cui ci si nutriva con con un intercalare piuttosto lungo nel tempo. Attualmente, con gli allevamenti intensivi e la produzione industriale, non ci ritroviamo più il gallo, la gallina e il maiale, ma ci ritroviamo banalmente delle vaschette di plastica coperte da un con all'interno un pezzo di un qualcosa che non necessariamente sappiamo da dove arriva. Visto e considerato che è piuttosto comodo alimentarsi in questo modo, se ne fa un uso spropositato e anche controproducente per la nostra salute. In sostanza, quella che era la nostra tradizione alimentare e culinaria italiana è andata a farsi benedire, in conseguenza della produzione industriale e degli allevamenti intensivi, che mettono a disposizione una quantità eccessiva e a buon prezzo di un alimento dannoso per la salute se consumato consumato in misura eccessiva. L'ordine del giorno in esame, che non necessariamente vuol trovare giustificazione alla carne coltivata - non è questo il punto - prova a risalire alle ragioni che dicono: facciamo ricerca in questo senso, perché

promuovere una campagna alimentare educativa finalizzata a una riduzione del consumo di carne, volta al raggiungimento di un complessivo, equilibrato e non eccessivo apporto di proteine animali. Tutto questo andrebbe a favore di tante circostanze: intanto intanto la tutela della salute degli italiani, affinché non mangino troppa carne; la riduzione degli allevamenti intensivi; il ripristino dei terreni per lo stoccaggio di CO₂. Questa è la prima parte dell'ordine del giorno, che mi sembra condivisibile anche ai fini della salute. La seconda parte riguarda la verifica della possibilità di convertire in forestazione parte dei terreni agricoli destinati alla coltura di cereali per l'alimentazione degli animali detenuti negli allevamenti e, parallelamente, per ridurre la quantità di impianti

e fare in modo che a tale visibilità pubblica corrispondesse anche una coerenza pubblica delle affermazioni che si fanno in

Aula, dal ministro Lollobrigida, che l'Italia non ha paura della ricerca: sono parole sue. Il senatore De Carlo ha affermato che non c'è passaggio che vieta la ricerca in questo Ancora, il Ministro ha affermato che la ricerca per noi è un elemento cardine, in particolare se si tratta di ricerca pubblica.

avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, alle emissioni di CO₂

Caro: quando 260 Nazioni nel mondo legiferano andando in una determinata direzione e un'unica Nazione va nella direzione opposta, è probabile che si vada verso una transizione alimentare.

disegno di legge alcun passaggio che vieta la ricerca scientifica *(Applausi)* e poi, quando si parla di bandi di ricerca scientifica pubblici, del Ministero della salute, bocciate questo emendamento? Come è possibile?

e con grande fiducia. Io però mi rivolgo, attraverso di lei, anche alla maggioranza. Mi rivolgo con fiducia al ministro Lollobrigida. Signor Ministro, perché vieta la ricerca pubblica? Lei sta vietando la ricerca pubblica. Perché la vieta? Ci spieghi perché vieta

solo tranquillizzare il collega Mazzella. È vero, siamo coerenti: non abbiamo messo alcun divieto alla ricerca. Il Ministro è stato addirittura più esplicito e ha detto che quella ricerca andrà fatta

colleghi, a solo una settimana dall'approvazione in quest'Aula del disegno di legge che celebrava l'agricoltura contadina, la sua valorizzazione e il suo primato nell'economia nazionale e che ci ha visti votare convintamente per la sua approvazione, questo ulteriore provvedimento a tutela del nostro patrimonio enogastronomico nazionale non può che trovarci in piena sintonia. Un plauso sentito va, dunque, al ministro Lollobrigida per aver dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti di un tema di primaria importanza, a cui mai e poi mai nessuna deroga deve essere accordata. Mi riferisco, signora Presidente, al tema della salute animale e umana, che il provvedimento in discussione intende salvaguardare.

per quelli che lui stesso ha definito essere i primi ambientalisti, cioè gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori. Non possiamo che essere d'accordo, signor Ministro, e veramente grazie per aver sottolineato sempre, in ogni suo passaggio su questo testo e anche nella sua azione quotidiana, il fatto che la parola "qualità" coincida, per lei e per tutti noi, per questa maggioranza, con il nostro Paese, cioè con l'Italia. Vietare la produzione e l'immissione sul mercato italiano di alimenti sintetici, oggetti del provvedimento al nostro esame, non poteva che essere quindi la naturale conseguenza dell'azione di questo Governo di centrodestra. Un'azione fondata sul rispetto delle tradizioni italiane, sulla salvaguardia dell'economia nazionale, sul *made in Italy* e sulla sovranità alimentare, come recita appunto, e non a caso, il nome del Ministero che ha voluto promuovere questa iniziativa legislativa. Vede, Presidente, l'abbiamo detto a gran voce in quest'Aula solo pochi giorni fa: l'Italia è da sempre un Paese a vocazione agricola. L'agricoltura è un vero e proprio è un vero e proprio motore dell'Italia e del suo tessuto socio-economico; ma soprattutto per noi l'agricoltura è vita, è amore per la nostra terra ed è quindi garanzia di cibo sano e di qualità, non del *junk food* e del nutri-score. Ogni singola Regione italiana esprime più biodiversità della maggior parte degli altri Paesi al mondo. Questo si traduce in una cucina italiana che valorizza i prodotti tipici dei territori regionali, una cucina considerata il nostro ambasciatore nel mondo e candidata come patrimonio UNESCO. In quest'ottica il cibo sintetico va nella direzione opposta a quella che è la nostra vocazione di alimentazione. Lo dico - e il Ministro lo sa bene - da animalista, che evidentemente non ama gli allevamenti intensivi e che più che altro consiglia a lei, Ministro, di farsi sempre interprete della salvaguardia del benessere animale e del trattamento degli animali. Ma lei - e la ringrazio ancora una volta - oggi ha ben spiegato in quest'Aula, nella sua prolusione, che anche con il cibo sintetico, purtroppo, gli animali non vengono salvaguardati; lo sono di più con i nostri allevamenti. *(Applausi)*. La nostra alimentazione è basata invece sulla valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche nazionali, simbolo di alta qualità e identificative dei territori e delle tradizioni nazionali. Dare il via libera al cibo sintetico nel nostro Paese - il "cibo Frankenstein", come lo chiama spesso il Ministro e che condivido - significherebbe esporsi al rischio concreto che l'agricoltura venga ridimensionata, con ovvie conseguenze sulle aree interne e con il loro progressivo spopolamento, che è uno dei problemi del nostro Paese. Lo dico con tono accorato, venendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, dove proprio dell'agricoltura e della salvaguardia dell'ambiente si è fatto invece un pregio; è per questo che da noi lo spopolamento non avviene. non avviene. Il cibo sintetico finirebbe per costare di più in termini di sostenibilità ambientale, senza alcuna certezza di migliore salute e nutrizione per i cittadini. Viene allora spontaneo chiedersi: *cui prodest*? Lo ha spiegato bene il Ministro poc'anzi: *prodest* agli investitori privati e alle multinazionali, che evidentemente non hanno lo stesso accorato interesse per i cittadini che possiamo avere noi, che siamo i legislatori pubblici. Se è vero, come è vero, che gli alimenti sintetici sono stati oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale, non solo in laboratorio, ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti, e se è vero, come è vero, che in alcuni Paesi extraeuropei addirittura sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione commerciale di tali alimenti e che negli Stati Uniti la Food and drug administration ha dato l'ok alla carne sintetica, ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio facendo sviluppare cellule animali, allora, onorevoli colleghi senatori, abbiamo di fronte un rischio non da poco. Ben presto si potrà arrivare ad una richiesta di commercializzazione di tali prodotti e di carne sintetica sul mercato europeo. Non a caso il rischio della diffusione di alimenti sintetici sul mercato europeo è cresciuto sensibilmente dopo il via libera da parte americana. Un rischio che questo Governo ha ritenuto di non dover correre, in assenza anche di una normativa europea comune sul tema, ritenendo al contrario che fosse quanto mai necessario procedere ad un'attenta valutazione prima della loro eventuale immissione sul mercato italiano. Infatti con questo disegno di legge viene sancito il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare cibi o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

non possiamo ignorare che da numerosi studi scientifici, ancora una volta condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, è emerso come solo poche ricerche abbiano affrontato, seppur brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. La ricerca e la sperimentazione degli alimenti sintetici sembrano quindi essere ancora in una fase embrionale tale per cui oggi non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, come è stato detto, di poter verificare quale sarà l'effetto

Al contrario, un consumo maggiore di alimenti ultralavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari e direi anche degenerative e anche questo purtroppo è scientificamente provato (e lo posso dire per esperienza Alla luce di tutto questo e, sottolineo, in assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, bene hanno fatto ancora una volta il Governo e il ministro Lollobrigida a intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale. Questo è il dovere dei legislatori italiani; questo è il dovere del Governo italiano, vale a dire, soprattutto, tutelare la salute dei cittadini. Se si dovesse imporre sui mercati la produzione di cibi sintetici, ci sarebbero maggiore disoccupazione, più rischi per la biodiversità e prodotti che, a nostro avviso, non garantirebbero Questo non significa avere un atteggiamento persecutorio, ma solo una forte volontà di tutela del patrimonio enogastronomico nazionale, della salute e del benessere umano, ma anche di quello animale che, come ho detto, a me sta particolarmente a cuore, quale diritto costituzionale. Il disegno di legge in esame va perciò nella giusta direzione, vale a dire quella di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana, degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il nostro patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale cui tutti in quest'Aula dovremo sempre badare e che tutti dovremo tenere nel cuore. Il nostro Paese, quale culla della tradizione agroalimentare mediterranea, deve continuare a promuovere stili di vita sani e stili alimentari naturali fondati sulla qualità e sulla tradizione. Un prodotto sintetico e ingegnerizzato non può sostituire la dieta mediterranea, non salva l'ambiente, perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute, perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare; inoltre, non è accessibile a tutti, poiché, come ho detto prima, è nelle mani di grandi multinazionali. A nostro avviso, basterebbero queste semplici ragioni a far propendere quest'Assemblea per un'approvazione unanime di questo provvedimento, che ha il merito di certificare, senza se e senza ma, la salvaguardia delle nostre produzioni nazionali nel settore zootecnico e della salute umana e animale, senza evitare qualsiasi tipo di sperimentazione, com'è stato detto, e di ricerca. Per tutte queste ragioni, signora Presidente, annuncio convintamente il sostegno del

oggi siamo qui a votare un provvedimento che, come ho già avuto modo di illustrare ieri in quest'Aula, appare nella sua illogicità immotivatamente contrario a qualsiasi avanzamento scientifico in tema di sostenibilità alimentare, ambientale, economica e sociale. È un provvedimento fazioso e - sì, lo ribadisco anche oggi - oscurantista, che rigetta *a priori* e senza alcun fondato motivo le istanze di innovazione e progresso che pure ci vengono suggerite a livello internazionale dalla comunità scientifica e dal mercato. Non volevo farlo, signor Presidente, ma mi sento chiamata in causa dal presidente De Carlo e dal ministro Lollobrigida, perché qui sta nascendo un grande malinteso. Lo ribadisco ancora: non sono gli agricoltori e gli allevatori ad essere retrogradi, per i quali anzi nutro e nutriamo la massima stima e rispetto; sono le politiche agricole e agroalimentari proibizionistiche e conservatrici ad esserlo, quelle messe in campo da questo Governo, che si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. politiche che stanno frenando il progresso comunque in atto. Parliamo di un settore di eccellenza composto da migliaia di piccole aziende, di cui andiamo orgogliosi, ad oggi costretto a fronteggiare, senza il concreto sostegno di questo Governo, sia le conseguenze derivanti dalla crisi climatica, sia le necessarie sfide

come si può definire questo disegno di legge, che con pregiudizio criminalizza la produzione e la commercializzazione di prodotti di cui il mercato italiano ancora non dispone? Amareggia e preoccupa la visione cupa ed eccessiva, offerta dalla maggioranza di Governo, circa i fantomatici rischi che il consumo della carne coltivata

il Governo Meloni è infatti abituato a cavalcare la paura del nuovo, dell'ignoto e del diverso, pur di portare avanti le proprie istanze conservatrici, che sono fuori tempo massimo. massimo. Il Governo, in palese difficoltà argomentative, invece di entrare nel merito, non si fa problemi a imbavagliare il diritto alla rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare o di stravolgerne le parole. Basti pensare anche solo all'utilizzo di una terminologia tendenziosa e scientificamente imprecisa: la scelta di utilizzare la dicitura "carne sintetica" e non quella corretta di "carne coltivata" è di per sé identificativo dell'opera di manipolazione operata da questo Esecutivo, volto a instillare nel consumatore l'impropria convinzione che la carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda nell'immaginario collettivo alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso alla salute. Ribadiamo, infatti, come i presupposti pericoli connessi alla sperimentazione di cibi a base cellulare, contrariamente alle tesi sostenute dalla maggioranza, non trovi alcun riscontro scientifico. Non c'è riscontro che supporti l'esistenza di problematiche specifiche di sicurezza alimentare derivanti dal consumo di carne a base di cellule coltivate. Tra i tanti *report* segnalo lo studio safety aspects of cell-based food*», compiuto dalla FAO e pubblicato a marzo 2023, ma non ci può essere, dato che la carne coltivata non è ancora in commercio. Diversamente, ciò non si può sostenere per la cosiddetta carne tradizionale, il cui abuso può essere causa di gravi patologie per l'organismo umano. Anche qui è bene sottolineare, differentemente da come siamo abituati a pensare, come il massivo consumo di carne convenzionale non sia nemmeno completamente ascrivibile al tradizionale modello alimentare italiano, come pure il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare si impegna a sostenere. Il consumo di carne, infatti, ha conosciuto una prima forte espansione solo a partire dagli anni Ottanta, per effetto della rivalutazione di modelli alimentari legati alla dieta mediterranea, dunque come conseguenza dell'affermazione di un comportamento consumistico differente dal passato. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra non mettiamo in discussione la sacrosanta esigenza di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano che ci contraddistingue e ci valorizza a livello internazionale e per i quali - ripeto - nutriamo massima stima e rispetto. Ciò che intendiamo esprimere in questo intervento è che la produzione della carne coltivata non minerebbe in alcun modo questo patrimonio. È infatti dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente distribuiti dalle virtuose aziende italiane. Insomma, aprendo all'opportunità di condurre studi sulla produzione di cibi a base di cellule coltivate, non saremo messi davanti a un atteggiamento del Governo di *aut-aut* quanto più di *et-et*. In questo modo, non solo si favorirebbe la nascita e lo sviluppo di un nuovo tipo di industria, più sostenibile e avente ricadute positive anche in termini di occupazione, ma al contempo si riconoscerebbe in capo al consumatore anche un più ampio diritto di scelta. Non è da sottovalutare infatti la percentuale di consumatori che ad oggi, per ragioni etiche, ambientali o anche strettamente sanitarie, potrebbe ragionevolmente intravedere in questi nuovi prodotti una valida alternativa alla carne convenzionale. Approvare oggi questo disegno di legge significa di fatto bloccare il progresso scientifico dell'Italia, rallentare il processo di transizione ecologica, privare di opportunità economiche le aziende e gli imprenditori che mirano a conquistare nuove fette di mercato, e non da ultimo generare attrito fra due fra due comparti: rispettivamente, quello dell'agricoltura tradizionale e quello futuro della carne coltivata, che coesistendo potrebbero costituire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema Aurora). Negare tutto questo preventivamente e unicamente sulla base di malferme intenzioni oscurantiste - lo ripeto, oscurantiste - non è certamente degno del Paese che siamo e che siamo chiamati a rappresentare. Per questo motivo, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, annuncio convintamente

già il titolo di questo provvedimento è pura propaganda. Prendete una possibile innovazione, la spogliate degli elementi di merito e la riempite di paure, con il solo scopo di presentarvi come quelli che proteggono i cittadini. Parlate di carne sintetica o addirittura di "carne Frankenstein", quando qui di sintetico non c'è nulla; anzi, si tratta di carne a tutti gli effetti. Addirittura portate il Parlamento a discutere del divieto di vendita di un qualcosa che non esiste, visto che in Europa al momento non c'è neppure una richiesta per autorizzare la carne coltivata, l'aggravante che quando nei prossimi anni l'EFSA ne autorizzerà il commercio l'Italia in ogni caso non potrà vietarne la vendita. Pertanto, più che eroi che salvano il Paese, ricordate Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento. Come se non bastasse, vietate per i prodotti vegetali di usare la denominazione dei tipici prodotti della carne. Questo quando tutti sanno che, per fermare il cambiamento climatico, si deve limitare il consumo e la produzione di carne. Vorrei ricordare che gli allevamenti intensivi impattano sull'ambiente con il 30 di suolo e circa l'8 per cento di acqua dolce, generando il 17 per cento di gas serra del pianeta. L'80 per cento degli antibiotici prodotti nel mondo servono per tenere in vita 5 miliardi di capi di bestiame di grossa taglia e 12 miliardi di polli e affini allevati nel mondo. Per non parlare delle enormi sofferenze di questi animali, che sono esseri senzienti, mentre invece sono ridotti a materiale per la produzione standardizzata agroalimentare: secondo tanti, è uno dei più grandi crimini commessi dall'umanità. Dite che vi fa senso la carne prodotta in un ambiente sterile, ma avete mai visto le immagini dei maiali negli allevamenti intensivi che per tutta la vita non riescono neppure a girarsi, dei conigli che non riescono a stendersi, delle mucche che per tutta la vita non vedono la luce del sole, dei vitelli trasportati per migliaia di chilometri fino in Nord Africa, dove vengono abbattuti secondo i riti locali? Tutto questo non vi fa senso? Dove sono gli animalisti del centrodestra che vanno sulle barricate per la vita di un orso o di un lupo e non dicono nulla su un prodotto che potrebbe salvare la vita di miliardi di animali?

Adesso all'orizzonte si prospetta una possibile soluzione che non comporta la sofferenza e l'uccisione di miliardi di esseri senzienti, che non consuma suolo,

Anche se è ancora in fase di sperimentazione, i benefici legati alla carne coltivata sono così importanti che provocheranno una rivoluzione nel nostro modo di mangiare e aiuteranno a sfamare un mondo che presto raggiungerà i 10 miliardi di abitanti. Voi invece cercate di fermare il futuro, ma la ricerca sulla carne coltivata andrà avanti in altri Paesi, incoraggiata e sostenuta dai Governi. Singapore, Stati Uniti, Israele e Olanda sono all'avanguardia di questa innovazione. Solo l'Italia rimane indietro. Eppure sulle cellule staminali e sulla produzione dei bioreattori è all'avanguardia e potrebbe diventare *leader* nella produzione di questo nuovo prodotto, visto che già oggi fornisce agli Stati Uniti e a Singapore la tecnologia per la produzione di carne coltivata. parlate di precauzione e di tutela del patrimonio agroalimentare, ma per la precauzione ci pensa l'EFSA, che ammette un cibo solo se è sicuro per la salute, così come succede con ogni medicinale. Poi non si capisce perché i protagonisti dell'eccellenza italiana alimentare dovrebbero temere la carne coltivata: è ovvio che non farà concorrenza alle produzioni di qualità. Poi non dimentichiamo che l'Italia importa il 50 per cento della carne che consuma. È proprio sullo sviluppo della qualità che dovrebbe concentrarsi il sostegno all'agroalimentare, il quale può essere solo avvantaggiato da un'alternativa a quegli allevamenti intensivi che riscaldano il pianeta, colpendo soprattutto le agricolture del Mediterraneo. colleghi, la vostra miopia infliggerà un danno immenso all'economia italiana. Nel mondo, le *startup* che lavorano sulla carne coltivata sono passate da 13 a 171 in soli sei anni ed entro il 2030 il giro d'affari potrebbe essere di 25 miliardi di dollari. Con il vostro *marketing* della paura fate perdere una grande opportunità, quella di produrre carne coltivata *made in Italy*. non dite che non vietate la ricerca, perché è chiaro che la fermate se vietate il possibile risultato. Signor Presidente, il provvedimento in esame è una mozione di sfiducia cinica e cruenta al mondo della ricerca e alla capacità del sistema agroalimentare di far crescere la sua qualità. Non si difende il *made in Italy* costruendo barriere sulla sabbia. Stavolta non siete i primi a fare qualcosa, ma l'unico Governo che prova a fermare il vento con le mani. E questo dovrebbe farvi riflettere.

ci sono due visioni diverse di cosa si può considerare allevamento *made in Italy*. C'è chi dice che bisogna andare verso la ricerca di nuove forme di produzione di cibo, perché in un mondo in cui aumentano le persone e aumentano i nuovi nati - non in Italia, non in Europa, non in Occidente, ma nel resto del mondo sì

che la natura deve venire prima di esperimenti futuribili, è sempre stato così nella storia del mondo; che la scienza deve venire incontro agli agricoltori, agli allevatori, per migliorare la qualità delle razze in oggetto, per migliorare la resistenza delle colture nei confronti dei cambiamenti climatici, ma che sempre di natura si deve parlare. Chi le parla ha un compito alquanto complicato, perché una parte del nostro Gruppo,

ma che si preveda un divieto preventivo alla vendita di alimenti di cui non si conosce ancora la portata. In seguito ad una ricerca Paese deve avvenire, perché noi siamo i migliori ricercatori, probabilmente si potrà anche cambiare idea. Perché, però, agiamo in anticipo? Perché siamo oscurantisti? Io penso ai 600.000 allevatori che, nel nostro Paese,

un allevatore, di cui non farò il nome perché non mi sembra corretto, nel farmi visitare con orgoglio la sua stalla, mi mostrava come al mattino venivano massaggiate e lavate, una per una, per garantire meno *stress* nella produzione di latte e maggiore qualità.

del mattino era un po' arrabbiato, ma era parte di un mondo in cui quella dimensione era tutto.

con un biodigestore, io produco una fettina, mi avrebbe guardato anche con un po' di fastidio. I suoi figli non fanno il mestiere dell'allevatore, perché è faticoso. L'ultima volta che sono stata nel mio collegio, quando l'ho invitato a venirmi a trovare lui mi ha detto che gli dispiaceva ma doveva produrre il fieno per l'allevamento. Erano le 7 di sera e lui era ancora lì. Io mi sentivo stanca perché faceva caldo e lui tutto il giorno era stato lì.

che io spero non arrivi mai. Lo spero per il mio amico Andrea, che con orgoglio mi ha aperto la forma di parmigiano alle 9 del mattino, facendomi prendere quattro chili e mezzo

quella carne non avrebbe gli stessi nutrimenti. L'abbiamo creata a nostra immagine e somiglianza, come possiamo pensare di creare a nostra immagine e somiglianza una bistecca 3D. Ma che gusto ha? Ha il gusto della mia carne piemontese? Ha il gusto della carne toscana, che è diversa? Ha il gusto della carne dell'alpeggio delle mie montagne: la transumanza, la bellezza di sentire il dondolio dei campanacci? Chi va a fare una passeggiata e vede le mucche, avendole sempre viste disegnate e mai naturali, quando le vede dice che sono qualcosa di bello? Che sapore avranno quei formaggi creati in laboratorio? Avranno il gusto della viola, della viola, quando riescono a mangiarla, e della lavanda? Perché adesso si fanno mangiare anche i fiori, in modo tale che i formaggi abbiano un sapore diverso. I 60 miliardi di *export*

Siamo proprio uguali agli olandesi, che creano quel formaggio giallo-arancione che non ha nessun sapore? Vantiamo sempre

il nostro olio, le nostre nocciole, la nostra crema spalmabile, anche quando non hanno il pane. In Cina la Ferrero vende tantissimi Ferrero Rocher, perché non avendo il pane non possono spalmare la Nutella, ma il cioccolatino che ha l'involucro dorato ai ricchi cinesi piace molto. Perché, allora, dire che quella bistecca fatta in laboratorio ha lo stesso valore di una vita di sacrifici e di come quelle che hanno i nostri allevatori e produttori? La ricerca ci deve essere. Personalmente, signor Ministro, sarei stata meno timida nell'accettare alcuni emendamenti che favorivano la ricerca, giusto per togliere gli alibi a chi oggi non voterà a favore di un provvedimento che va

la ricerca che oggi parla di futuro parli anche con quegli allevatori che hanno paura di perdere il posto di lavoro. Prima di prendere una posizione, tendenzialmente leggo sempre, proprio per evitare che i miei pregiudizi

Questo accordo, però, ha fatto sì che le arance marocchine invadessero i mercati di tutta Europa. Ovviamente i lavoratori in Marocco vengono pagati molto di meno e quindi veramente le arance marocchine, che vengono prodotte con meno attenzione rispetto a quelle siciliane, hanno invaso l'Europa e i nostri agricoltori siciliani hanno avuto un nocumento da un accordo che era nato per un fine positivo: evitare

di aprire la forma di formaggio e massaggia la mucca con l'acqua, perché penso che debba essere tutelato lui per primo. Poi, quando un giorno scopriremo che tutta questa carne è carne e che non arreca danni alla salute, lasceremo che il consumatore, dopo essere stato informato, scelga se salvare Andrea Andrea o salvare un laboratorio chimico; sarà la scelta del consumatore, per oggi io salvo Andrea.

questo è il nostro Paese, un Paese in cui si mangia. In discussione non c'è solo il tema della nutrizione, che chiaramente non può essere sottovalutato, tuttavia si dice che in molti Paesi del mondo mentre in Italia il mangiare ha a che fare con la cultura, con la famiglia, con i valori. Questo non possiamo negarlo, dobbiamo portarlo avanti, riconoscerlo e conservarlo, perché fa parte del patrimonio del nostro Paese. Con il disegno di legge in esame il Governo propone proprio di tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, perché rappresenta la nostra società, la nostra cultura, la nostra economia,

a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, cioè i mangimi sintetici. Chi non è intimorito anche da questi termini? Abbiamo infatti a che fare con un futuro che dobbiamo affrontare (perché dobbiamo farlo), tuttavia che la carne sintetica venga prodotta attraverso un procedimento biotecnologico, estraendo e poi lavorando cellule staminali da animali adulti o da embrioni di animali

stato poi introdotto il divieto di utilizzare la denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, così come quello di utilizzare nomi che fanno riferimento alle specie animali, alla loro morfologia o anatomia. Allo stesso modo non potranno essere utilizzati nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali, questo perché

No, l'Italia rimane avanti, dove è e dove vuole restare, con la qualità dei propri prodotti, dei propri allevamenti, del proprio cibo e del proprio patrimonio culturale ed enogastronomico. Non confondiamo il tema della ricerca, alla quale siamo favorevoli, con quella parificazione e confusione alla quale diciamo di no alla quale diciamo di no con chiarezza. È vero che bisogna dare da mangiare a tutti, però dobbiamo anche spiegare a tutti che le tradizioni, che fanno parte di un patrimonio di centinaia di anni, non possono essere cancellate. Io vengo da una provincia in cui lo spiedo bresciano è intoccabile; le peppole e i fringuelli fanno parte della vita di più generazioni e ancora facciamo fatica a spiegare perché non possiamo più consumarle, ma in cambio alcuni in Europa ci dicono che possiamo mangiare le cavallette e gli insetti. Questa cosa ancora non l'abbiamo capita, non la digeriamo e non la digeriremo mai. anche in questa direzione dobbiamo andare, perché possano essere tutelate le nostre origini e le nostre tradizioni. E allora va bene che siano definite le autorità preposte ai controlli e che siano previste le sanzioni e le modalità per applicarle ai produttori che trasgrediscono. trasgrediscono. Apro una piccola parentesi. Nessuna intenzione di mettere all'indice vegetariani o vegani, posto che ciascuno fa le scelte dietetiche e salutistiche che ritiene più opportune.

Significa anche dare una più puntuale riconoscibilità ai prodotti alimentari che andiamo ad acquistare. Questo vale per tutti, come diceva la collega che mi ha preceduto. In un futuro, quando ci sarà anche la carne artificiale, sarà la scelta di ciascuno che indirizzerà i consumi, ma nella chiarezza, nella trasparenza e nella conoscibilità, non nella confusione o addirittura nella parificazione, perché pari non sono questi prodotti. Questa riconoscibilità, che deve essere data ai prodotti alimentari che andremo ad acquistare e a consumare e che i nostri figli andranno a consumare, deve essere fatta adeguatamente. I vegetariani potranno continuare ad acquistare i prodotti, stando attenti a seguire le denominazioni che verranno date dai produttori di questi alimenti, ci mancherebbe. Ma bene fa il Governo - e noi sosteniamo questa azione - a tutelare la carne e i suoi produttori. Salvaguardiamo i produttori italiani, affinché producano e continuino a produrre carni sempre migliori e di qualità, ricordando le raccomandazioni di chi (la ricerca ed altri) ci invita a un consumo non eccessivo di carne animale, ci mancherebbe. Ma, allo stesso tempo, certamente non demonizziamo chi cerca in altri alimenti le proteine e le vitamine così importanti per la nostra alimentazione.

pleonastico, inutile o eccesivo. Non è vero. Noi vogliamo dire chiaramente ai nostri produttori che li difendiamo e vogliamo dire chiaramente ai nostri concittadini che difendiamo la chiarezza e l'origine dei consumi alimentari nel nostro Paese, difendiamo quella tradizione che permette

e della *ratio* dell'insieme di queste norme che il Governo ha messo in atto, quindi voteremo a favore del disegno di legge al Signora Presidente, quasi mi dispiace dover interrompere questo clima idilliaco che si è creato tra la maggioranza e una parte della cosiddetta opposizione. Ministro, un po' di realtà, purtroppo, anche a dispetto della sua lunga e devo dire appassionata requisitoria, va riportata in quest'Aula, perché rimane un dato di fatto: questo provvedimento rappresenta davvero un oltraggio al Paese e a questo Parlamento, che è stato tenuto impegnato per settimane a lavorare su un testo bandiera, forse il peggiore tra quelli prodotti finora dall'insediamento di questo Governo, a partire dal famigerato decreto *rave*. Si tratta di un manifesto di ignoranza intriso di malafede, Ministro, io non credo che alla sua intelligenza questo sfugga. Lascia davvero attoniti il fatto che un Governo, che dovrebbe difendere i propri cittadini dalle *fake news* si faccia invece promotore di *fake news* *(Applausi)* e contribuisca quindi ad alimentare quel clima complottista che sempre più purtroppo in Italia impedisce un dibattito sereno e serio sugli argomenti. State vietando, infatti, ciò che ancora non esiste, ma che tutti i dati ci dicono che potenzialmente diventerà una fetta enorme del mercato italiano, internazionale e mondiale. dunque a fare un po' di chiarezza, perché avete anche scelto deliberatamente di utilizzare termini scientificamente scorretti e quindi falsi, che inducono in errore. Proviamo a capire di che cosa parliamo. Stiamo parlando del processo produttivo della *cultivated meat*, la carne coltivata, che prevede la coltura di cellule isolate a partire da una piccola parte prelevata da un animale vivo, tramite prelievo di sangue o biopsia effettuata in anestesia locale, senza necessità di macellazione dell'animale stesso. Dal materiale ottenuto dal campione si isolano le cellule staminali e si ricreano in situazioni controllate le condizioni di crescita che fisiologicamente le cellule avrebbero all'interno del corpo dell'animale. Una volta ottenuto il quantitativo adeguato di cellule, esse sono lasciate maturare perché possano sviluppare e differenziarsi in cellule muscolari, in tessuto adiposo, in tessuto connettivo. Le quattro fasi del processo produttivo della carne colturale, come indicato dalla ricerca della FAO e dell'OMS citata anche in quest'Aula e pubblicata a marzo 2023, sono rappresentate dall'approvvigionamento delle cellule, dalla produzione, dalla raccolta e dal trattamento alimentare. Questo è il processo che viene definito come agricoltura cellulare e le cellule vengono coltivate in un brodo ricco di nutrienti necessari a facilitarne la proliferazione. Questo brodo non contiene qualche sostanza magica o chimica o chissà che cosa, ma contiene acqua, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali. La carne coltivata, ciò di cui stiamo parlando oggi, esiste attualmente in Europa solo a livello sperimentale, come lei sa bene, Ministro, mentre è già in commercio soltanto in USA, Singapore e in Israele. Si prevede, però, che l'introduzione sul mercato internazionale avverrà sì gradualmente, ma molto velocemente e sarà già disponibile su larga scala nel 2030. La carne colturale è la sfida scientifica del prossimo decennio, quella sfida che con questo divieto preventivo, che voi istituite, state facendo perdere all'Italia. *(Applausi)*. Altro che difesa degli interessi della Nazione. È vero che è ancora in fase sperimentale, ma alcune stime sul suo potenziale esistono già, sono fornite dalla Mosa Meat, ma anche da nostri ricercatori, ricercatori italiani dell'università di Trento. Tali stime dicono che sono necessarie tra le due e le dieci settimane per ottenere un prodotto cellulare completo e, poiché la crescita delle cellule è esponenziale, da un singolo ciclo produttivo sarà possibile coltivare 100.000 *hamburger*.

di carne di manzo: ciò significa che stiamo guardando ad una potenziale prospettiva per cui, prelevando dei campioni di cellule da sole 150 mucche, si potrà soddisfare l'intera attuale domanda di carne. Questo è il mercato potenziale cui si sta guardando. Quest'anno ci sono 156 *startup* mappate; soltanto nel 2021 erano 107. Anche questo indica una grossa crescita di questo settore. In Italia c'è una sola *startup* che si occupa di coltura cellulare, la Bruno Cell, che nel 2021 ha partecipato, insieme a un'azienda statunitense, a un bando dell'ESA, l'Agenzia spaziale europea,

di avere un costo affrontabile per trasportare le derrate alimentari e avere la possibilità di coltivarle *in situ* è qualcosa cui il settore aerospaziale sta guardando, un altro settore dal quale state coscientemente tagliando fuori l'Italia, nuovamente alla faccia dei patrioti. Però, Ministro, c'è molto di più: io l'ho sentita addirittura parlare di volontà popolare. Allora, mi consenta, perché è chiaro che lei faceva riferimento a quella famosa petizione quella famosa petizione di soggetti direttamente interessati ad impedire lo sviluppo di questo settore. Ebbene, quella famosa petizione ha raccolto - sì - circa mezzo milione di firme, che però rappresentano il 30 per cento dei loro iscritti e lo 0,8 per cento della popolazione italiana. Quello che lei ha fatto e questo Governo ha fatto non è stato ascoltare la volontà popolare, ma è stata un'azione lobbistica istituzionale. Nient'altro che un'azione lobbistica istituzionale a danno di quelli che sono i veri interessi del futuro di questo Paese. Ancora, questo provvedimento illiberale rischia di essere anche incostituzionale per due ragioni: per la violazione dell'articolo 9 e per la violazione dell'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 9 della nostra Costituzione, comma 1, dice che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Ho sentito sia lei, Ministro, che il presidente De Carlo affermare, a ragione, che in questo provvedimento non c'è alcun divieto di ricerca, ma se voi impedite - come fate con come fate con questo provvedimento - qualunque interesse di investitori pubblici e privati ad investire in questo tipo di ricerca, perché non c'è sbocco e non c'è il mercato per i prodotti di questa ricerca, voi la state soffocando. Quindi, affermare che non c'è il divieto, significa ancora una volta prendere in giro noi e anche i vostri elettori.

Ora è evidente che questo provvedimento sta invece stroncando l'iniziativa economica privata sulla base di un pregiudizio, perché non c'è alcuna dimostrazione scientifica che questo prodotto sia dannoso alla salute. Noi sappiamo che l'articolo 41 prevede che l'impresa privata è libera, purché non danneggi la salute e l'ambiente. Voi non potete affermare che lo faccia, quindi di fatto state impedendo la libera impresa nel nostro Paese. Ancora, ciò che si sa di questo possibile prodotto è, anzi, che possa far bene all'ambiente, all'ambiente, alla salute umana e al benessere degli animali; tutti gli indicatori vanno da questa parte e non il contrario, come affermate voi. Vedete, Vedete, la vostra tattica ormai la conosciamo molto bene: voi accusate gli altri di essere ideologici, mentre non c'è nulla di più ideologico di questo divieto che ha ribadisco - il suo unico fondamento in una politica di stampo "di interesse di pochi", perseguita in maniera metodica da questo Governo, a danno dei molti. C'è un'altra verità che noi e anche voi conosciamo molto bene ed è che il settore zootecnico nazionale è responsabile del 70 per cento di tutte le emissioni derivanti dal settore agroalimentare

630 milioni di animali. Se voi pensate veramente che questo sia un sistema alimentare sostenibile significa che non avete presente davvero quali sono i dati reali. Mi avvio alle conclusioni.

Questa maggioranza è forse all'avanguardia, ma è all'avanguardia della retroguardia. Prendete in giro i vostri elettori promettendo di poter far tornare il mondo indietro a prima della rivoluzione tecnologica e a prima della rivoluzione industriale; probabilmente, ispirandovi ai vostri valori, vorreste tornare indietro anche a prima della Rivoluzione francese, prima che fosse sancita l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e fossero definiti i diritti universali della persona. *(Applausi)*. terminare, ma questo è davvero importante per definire la cifra di questo provvedimento - che i consumatori vanno tutelati e non truffati, quindi volete imporre un vocabolario vietando l'utilizzo di alcune parole e segnatamente quelle che si riferirebbero a prodotti di carne e che non possono essere usati invece per prodotti a base vegetale. Vietare delle parole viene fatto soltanto in sistemi dittatoriali e retrogradi *(Applausi)*; non viene fatto nelle democrazie avanzate. Questa è follia. Aggiungo come nota quasi personale che bevo latte sintetico da venticinque anni, mi nutro di bistecche a base vegetale da quindici, e le mie analisi, facendo i dovuti scongiuri, sono perfette. Quindi mentite sapendo di mentire. Voglio chiudere con un ringraziamento alla Lega antivivisezione italiana (LAV), alla Bruno Cell, ossia l'unica *startup* in Italia che sta studiando il processo di produzione della carne coltivata, e ai tanti, tanti docenti universitari che stanno dando il loro contributo perché, al di là

*(Applausi)*, gli italiani possano accedere a fatti e dati reali. Il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, voterà decisamente contro questa vostra vergogna.

che espone il nostro Paese a un rischio eccezionale e mai visto prima. Noi siamo in trincea e dobbiamo difendere in ogni modo la salute degli italiani e la nostra economia. Ricordo a chi non conosceva i numeri prima di oggi che la filiera zootecnica italiana vale 55 miliardi di euro e conta un totale di 550.000 addetti; non ci sono solo animali macellati, ma anche addetti che - lo Tutto questo viene messo a rischio da carne, latte e pesce sintetici. Ricordo che, secondo un sondaggio Censis, l'84 per cento degli italiani si è dichiarato contrario all'idea di cibi prodotti in laboratorio: dalla carne, al latte, ai formaggi, al pesce. al pesce. Ma il rischio esiste ed è alto, tant'è vero che recentemente la Food and drug administration americana ha sdoganato i polli sintetici, e l'EFSA potrebbe anche autorizzare entro la fine dell'anno in Europa i cibi prodotti dalla clonazione di cellule staminali. Inoltre, in Danimarca si sta introducendo il latte sintetico e in Germania sono pronti i pesci e il sushi realizzati in laboratorio. Il *made in Italy* a tavola, messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico, vale quasi quasi un quarto del prodotto interno lordo nazionale: 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, 330.000 realtà della ristorazione, 230.000 punti vendita al dettaglio e 10.000 agricoltori impegnati in Campagna Amica con la vendita diretta. Per questo motivo condivido totalmente lo scopo del provvedimento fortemente voluto da questo Governo.

vogliamo dichiarare l'Italia come la prima Nazione libera dal cibo sintetico, intervenendo precauzionalmente a livello nazionale per tutelare gli interessi legati alla salute delle persone e al patrimonio gastronomico e agroalimentare del nostro Paese. Ne sappiamo ancora troppo poco e lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di questi alimenti sintetici. Lo scopo di questo disegno di legge sta tutto nell'articolo 2, che stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare e distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, in base al quale, se viene individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio. Il provvedimento prevede anche sanzioni amministrative per chi viola questi divieti.

ulteriore artificio utilizzato per avallare e diffondere l'impostazione che si sta facendo sempre più strada, cioè quella di confondere e ingannare i cittadini e dar loro l'impressione che finto equivalga a vero, convincendoli che stiano acquistando prodotti che contengono anche proteine di origine animale, quando invece non è così. Di conseguenza, gli italiani non troveranno più sugli scaffali dei nostri supermercati etichette con nomi fuorvianti, come bistecca di soia o di *tofu*, *hamburger veg*, mortadella vegana o altro. Con questa modifica si vieta infatti l'utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati, per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali. Con il nostro emendamento vogliamo assicurare il diritto ad una informazione corretta dei cittadini, per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma riconosciamo e difendiamo anche il valore culturale, socio-economico e ambientale dei nostri prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Siamo convinti infatti che chi vende prodotti con etichette ambigue compie una concorrenza sleale e anche per questo, con la nuova norma, rischierà pesanti sanzioni.

vegetale sono ricavati da materie agricole comuni, come i legumi, i cereali, i semi o le verdure, o dalle loro proteine isolate. Sono prodotti con ingredienti ritenuti unanimemente sicuri da tutte le autorità preposte alla sicurezza alimentare e che nulla hanno a che fare con i cibi sintetici, da laboratorio o da insetti. Perciò tuteliamo questi prodotti, ma un'etichettatura corretta può salvare il tutto. I cibi sintetici, poi, non sono cibi, ma sono "prodotti Frankenstein", ingegnerizzati e realizzati con processi più simili a quelli di produzione dei farmaci e come tali devono essere valutati e sottoposti quindi al medesimo processo di verifica, molto più approfondito di quello del *novel food*.

Una ricerca dell'università della California ha infatti elaborato un dato statistico, secondo cui la carne sintetica produce una quantità di anidride carbonica, emessa per ogni chilogrammo prodotto, da 4 a 25 volte superiore alla carne bovina tradizionale. Inoltre la carne coltivata non solo emette più CO2, ma consuma anche più acqua, come è stato detto in precedenza, e usa più combustibili. Viene quindi da chiedersi perché l'Europa e anche una parte dei parlamentari del nostro Paese spingono così tanto sulla carne sintetica.

e via via si estenderà a molte altre produzioni, che difendiamo con la nostra sovranità produttiva. Addirittura nei giorni scorsi abbiamo assistito a Facebook che ha bloccato la campagna informativa di chi parlava contro il cibo sintetico, dicendo che doveva utilizzare il termine "carne coltivata". Il secondo motivo è che questo tipo di produzioni rientra in una filosofia che è più vicina alla cultura angloamericana. C'è un abisso tra i sistemi di valori legati al cibo, come ha detto bene prima il Ministro: da una parte, quello dei Paesi mediterranei, Italia in testa, dove il cibo fa parte della cultura nazionale: è una tradizione, un'identità, un piacere da condividere a tavola. Al contrario, nei Paesi anglosassoni il cibo è considerato esclusivamente per la sua utilità.

genuino. Ecco perché ho iniziato il discorso affermando che il nostro Paese è in trincea, una trincea che va difesa dalle follie dell'Unione europea e dall'attacco dei grandi interessi che mirano solo al profitto. Dobbiamo difendere il benessere dei cittadini e la nostra economia, di cui l'agroalimentare rappresenta una fetta importante, ma anche la nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, che altrimenti non verrà più difesa. A questo proposito, voglio citare Ippocrate: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. È tutto qui. Noi siamo di fronte a un bivio. Conosciamo i benefici della dieta mediterranea, del cibo vero, del cibo naturale, la medicina che da millenni si prende cura di noi italiani, mentre non siamo certo sicuri degli effetti del cibo sintetico. Allora sia chiaro che noi scegliamo la dieta mediterranea, perché questo è il nostro cibo. Ciò che deve indirizzare l'azione di chi siede in queste aule è la tutela del benessere della popolazione italiana e credo sia chiara la scelta che noi siamo chiamati a compiere. Ebbene, per la difesa della nostra cultura e delle tradizioni di tutti i cittadini italiani,

Il decreto-legge in esame, oggi rinominato in virtù anche di un emendamento proposto dal Partito Democratico ed approvato in Commissione, fa sì che noi abbiamo una riformulazione puntuale. puntuale. Il modello che noi vogliamo è la definizione esatta di ciò che facciamo, con una corretta definizione, non solo terminologica, ma che si deve riportare anche su tutte le etichette che definiscono le caratteristiche del prodotto.

Oggi più che mai, a fronte di una serie di fattori inerenti ad una più marcata globalizzazione del mercato, sia per quanto attiene alla vendita che alla produzione, si impone sempre con maggior forza, l'esigenza di migliorare il percorso della trasparenza sull'origine del prodotto, le sue qualità, i metodi di produzione, la sostenibilità, affinché ci sia la dovuta chiarezza e consapevolezza da parte del consumatore. Questo è uno strumento di valorizzazione dei nostri prodotti, perché i consumatori possono scegliere e scegliere consapevolmente ciò che sono chiamati a consumare. Un principio, questo, che è condiviso dalle imprese e dai consumatori, che dimostrano una sempre maggiore, più attenta e crescente attenzione verso le filiere corte, alla qualità della produzione e alla sostenibilità ambientale. Il termine sostenibilità lo useremo spesso, perché è un elemento che dà valore ai prodotti e non è alternativo al prodotto stesso. Si condivide il principio ricorrente di chi, giustamente, ritiene che l'attenzione agli aspetti immateriali del rapporto con il cibo, alle persone che ci sono dietro e che ci mettono la faccia, il lavoro e la fatica, alle caratteristiche organolettiche, all'equità della distribuzione dei margini economici lungo la filiera, ai territori e al rispetto degli ecosistemi, siano tutti aspetti ormai divenuti intrinseci nell'alimentazione umana in quanto tale. Da qui non si torna indietro. Essi rappresentano valori condivisi dalla società in generale e non più la riserva simbolica di una nicchia ristretta di consumatori. Queste parole sono mutuate dal mondo agricolo, ma le facciamo nostre e credo che siano la luce e la via che dobbiamo perseguire nell'assunzione dei nostri provvedimenti. Tutto ciò, del pari, non deve però comportare una diminuzione degli *standard* in materia di sicurezza alimentare e dei soggetti chiamati a garantirla. In questa materia, un ruolo fondamentale lo riveste l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non ci si può sostituire a quest'autorità, a questi strumenti di controllo. Nella fattispecie, ancora nessun *dossier* per la carne coltivata è stato depositato presso detto ente. La nostra posizione - lo voglio chiarire a nome del Gruppo - non è equivoca, ma è chiara e indiscussa ed è allineata anche con quella dei nostri amministratori, che condividono la *ratio* della norma. *(Applausi)*. È la *ratio* indicata in tutti gli atti che sono passati dalle Commissioni, è quella di sostegno alle produzioni locali, di filiera, tradizionali e sostenibili, le quali rappresentano la nostra storia, la cultura, la cucina, la tradizione dei nostri territori, i quali molto spesso, come già detto da altri, sono conosciuti nel mondo non solo per le bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, ma anche per le loro produzioni. Tutto questo, però, non si contrappone a un'idea di futuro, di modernità dell'agricoltura e anche di evoluzione merceologica. Questo è il tema su cui spingere per valorizzare le produzioni, cioè far crescere la qualità e la sostenibilità della nostra agricoltura nella modernizzazione; le produzioni devono essere remunerate con il giusto prezzo per le imprese e per i lavoratori. Ci dev'essere una marginalità, oggi messa sempre più in discussione anche dall'andamento delle produzioni, conseguente ai cambiamenti climatici.

che fanno sì che un simbolo, un valore, un prodotto e un fatturato siano veramente messi a rischio. Ma com'è nato tutto questo? È nato di valorizzare le nostre denominazioni di origine, che sono circa 850. Sono circa 300 i consorzi, nati decine di anni fa da persone che non avevano nemmeno una formazione culturale, ma che sentivano l'esigenza di stare insieme per valorizzare questi prodotti. con la loro unità di intenti, hanno portato avanti quella qualità, quell'idea, quel sogno che hanno fatto bene alle loro attività, ma hanno fatto bene anche ai nostri territori e oggi fanno sì che possiamo dire di essere fieri del nostro *made in Italy.* migliorare la filiera e molte sono le azioni da compiere, che elencherei, senza dover dettare la linea, ma solo a titolo di contributo: bisogna agire sulla cultura della nutrizione e del benessere alimentare, con un'educazione alimentare anche nelle scuole nelle mense delle scuole, come avviene in molti Comuni, che vanno incentivati; bisogna operare sulla normativa, affinché sia rispettosa della trasparenza e della corretta informazione; bisogna operare sulla valorizzazione e promozione territoriale dei consorzi, perché ci sia sempre maggiore integrazione tra prodotto, territorio e cultura; bisogna esplorare i nuovi mercati e l'*e-commerce*, che ha salvato i nostri produttori anche nel periodo del Covid. Per fare tutto questo, però, bisogna mettere a punto un piano infrastrutturale potente da calare sui territori, affinché tutte le imprese agricole siano messe nelle condizioni di dialogare con il mondo e non siano isolate e confinate all'interno dei loro poderi. Questo è un tema che solleviamo tutte le volte, è un tema di competitività che necessita delle risposte che noi speriamo possano essere date. Bisogna lavorare sull'ammodernamento delle imprese agricole, sull'agricoltura di precisione e anche sulla ricerca. Il miglioramento passa dalla transizione ecologica, che migliori il benessere animale e favorisca gli allevamenti estensivi e l'agricoltura di qualità, che attiene molto alla ricerca e alla gestione delle immissioni. Ci sono molte *startup* che stanno anche avendo risultati innovativi e promettenti e vanno sostenute. Bisogna ridurre lo spreco del riuso delle acque reflue e non; bisogna sviluppare e migliorare le varietà, nel rispetto dell'autonomia varietale. Questo sarà un tema essenziale, perché dal miglioramento della resistenza idrica e dalla malattia delle varietà passeranno molte delle nostre sfide conseguenti anche alla necessità di adeguarsi ai cambiamenti climatici, che stanno creando condizioni spesso a noi sconosciute e che mettono in difficoltà i nostri agricoltori. Bisogna passare dall'efficientamento delle aziende (è positivo il provvedimento sull'agrivoltaico), ma con dei limiti, perché non sia lo strumento per il consumo del suolo e la cementificazione dei suoli e non metta in discussione le scelte che i territori hanno fatto venti o trent'anni fa, quando hanno deciso di vivere la loro ruralità, il loro paesaggio, la loro storia e la loro cultura. Che non si acceda a queste misure per fare speculazione energetica, perché questo non sarà ammesso e non sarà possibile. Bisogna valorizzare la biodiversità produttiva, valorizzando anche i settori che talvolta sembrano essere minori. Penso al tema degli impollinatori, magari residuale, ma essenziale per la vita dei nostri territori e delle nostre produzioni. al tema della ricerca meccanica e gestionale per l'agricoltura di precisione, al tema della ricerca nella medicina veterinaria e al tema dello sviluppo e della ricerca nel settore dei prodotti fitosanitari e degli erbicidi: quando la ricerca supererà gli attuali erbicidi (parliamo del glifosato e di altri), rispetto ai quali sappiamo tutti che sono in campo autorevoli ricercatori e moltissime risorse, potremo dire che potremo cambiare l'agricoltura e che andremo verso un'agricoltura più sostenibile anche nell'ambito biologico.

Pensando sempre di andare dritti senza mai volgere la testa a destra o a sinistra, a volte si rischia di prendere una strada che poi non porta il risultato sperato. Noi siamo stati collaborativi sul disegno di legge sull'agricoltore custode, perché ci crediamo: è quello il metodo di affrontare le questioni e le discussioni.

L'agricoltura si deve avvalere anche di un piano di gestione faunistica, non distinguendo tra l'agricoltore e chi gestisce il sistema faunistico venatorio. Intendo dire che un sistema marcia bene se marcia unito, se non ci si divide e se sui provvedimenti talvolta ci si ferma, si fa un po' di chiarezza rispetto agli equivoci e

esprimo quindi un voto di astensione, con la consapevolezza che un percorso potrà essere fatto, perché comunque la nostra agricoltura sia sostenuta, valorizzata nella sua storia, nella sua cultura, nella sua tradizione, nella sua biodiversità e nel valore che ci ha fatto dire di essere orgogliosi di essere orgogliosi del *made in Italy,* grazie al lavoro delle donne e degli uomini che nel tempo ci hanno creduto e di cui oggi siamo beneficiari e dobbiamo essere custodi.

la polemica, ovviamente, fa parte del Parlamento e della discussione, quindi questa Presidenza ne è garante. Parlarsi però singolarmente o, in un qualche modo,

la *vis* per introdurre la giusta polemica ed emozione nel suo intervento. La prego di continuare e la ringrazio anche. Grazie, Presidente, perché posso continuare. Vorrei spiegare il motivo del mio ringraziamento. Il problema per noi della maggioranza, collega Maiorino, è che, condividendo molto spesso *in toto* i provvedimenti che vengono dal nostro Governo, come questo, si perde l'energia necessaria per sostenere il dibattito in Aula, condividendo completamente il provvedimento. Ci viene quindi naturale considerare poi scontato il nostro intervento in Aula. I suoi interventi invece,

parlare. Si rivolga alla Presidenza e vedrà che tutto procederà benissimo. dell'aggettivazione esasperata negli interventi che ho ascoltato: posso citare "oscurantisti contro il progresso", posso citarlo, sì?

"un testo di ignoranza istituzionale" e, in chiusura della dichiarazione di voto, "il MoVimento 5 Stelle voterà contro questa vergogna".

Queste affermazioni sono però uscite dall'opposizione, non dai banchi della maggioranza e tanto meno dai banchi di Fratelli d'Italia. Quando io ringrazio, lo faccio sentitamente, perché ci dà modo, come maggioranza, di trovare gli argomenti e l'energia necessaria per sostenere il dibattito d'Aula. Quindi grazie di esistere, dicevo. Ora, per riportare un attimino il dibattito sul necessario livello di cultura,

è un protocollo di produzione di carne cosiddetta sintetica, o anche detta carne coltivata, perché consiste in una coltura cellulare che inizia con il prelievo di cellule muscolari e muscolari e di fibroblasti da un animale vivo. Le cellule vengono fatte crescere per selezionare quelle più adatte a proliferare in cellule staminali, ovvero cellule che hanno una grande capacità di proliferazione e di trasformazione in tipi differenti di cellule, quali quelle muscolari. Per farle crescere, le si alimenta con un mezzo nutritivo, che è il siero fetale bovino, molto prezioso, in quanto contiene fattori di crescita, ormoni e chelanti. Va sottolineato che l'uso del siero fetale di vitello, passaggio chiave per la produzione industriale di questo protocollo, non è sicuramente un metodo *cruelty free*, cioè non è indolore per la sua estrazione, né rassicura sul rischio di trasmissione di malattie come quelle da prioni, impossibili da diagnosticarsi in vita. si aggiungono amminoacidi, acidi grassi, zucchero, oligoalimenti e sali. Nelle diverse fasi di coltivazione, vengono aggiunti tripsina di maiale, nonché antibiotici e antimicotici, allo scopo di prevenire contaminazioni batteriche e fungine. Infine, per raggiungere l'immortalizzazione delle cellule di pollo perché questo protocollo attiene alla produzione di carne di pollo - viene introdotto un cisgene, cioè un gene negativo che fa parte del corredo genetico del donatore. È evidente che siamo di fronte a un cibo molto processato, un "cibo Frankenstein", come ha detto un nostro collega, per la presenza di numerosi farmaci e additivi, la partecipazione di tre specie animali e, infine, l'introduzione di un gene. Nel momento della lavorazione industriale è plausibile che il prodotto andrebbe a complicarsi ulteriormente, con la necessità di utilizzare diversi additivi per conseguirne il gusto e l'aspetto desiderati. I diversi passaggi evidenziano che possibili contaminazioni da parte di virus e batteri provenienti dalle fonti animali di origine oppure ambientali su un prodotto sintetico riprodotto in larga scala potrebbero ampliarsi a quantità impressionanti.

come nuovo cibo, perché è in realtà più un farmaco che un cibo: non a caso, il testo di legge è firmato dal nostro Ministro dell'agricoltura e dal nostro Ministro della salute. Il principio di precauzione che ho sentito più volte evocare ci induce a raccontare correttamente questa formula di produzione e a rivendicare ad oggi - e qui tranquillizzo anche rispetto ad alcune affermazioni che venivano

Quindi sì, è un testo bandiera; sì, è la nostra bandiera, che fa chiarezza rispetto a quello che reputiamo giusto - e su cui investiamo le istituzioni parlamentari per decidere sui provvedimenti adatti - e quello che reputiamo sbagliato.

autorevoli esponenti dei Verdi, come ad esempio, uno per tutti, Carlo Ripa di Meana, che fece un'autentica battaglia di vita contro gli OGM, perché giustamente difendeva le produzioni nazionali e la nostra capacità di stare nella nostra natura e nei nostri schemi di alimentazione.

Io non lo reputo un progresso: un protocollo di produzione come quello che vi ho letto, che - lo ricordo - è l'unico oggi approvato dagli organismi regolatori mondiali, cioè la Food and drug administration, non non è progresso, ma alta tecnologia alimentare; è ingegnerizzazione del cibo. Non ci appartiene o, quantomeno, non ci appartiene oggi, in questo momento storico. Non so domani quello che accadrà. Questa è una legge: se il progresso - che voi definite tale - veramente progredisce su percorsi maggiormente rassicuranti, che che rispecchiano il principio di cautela, come per tutte le leggi essa sarà in quel momento riconsiderata e riaffrontata, ma ad oggi il quadro che ci si presenta è questo ed è altamente preoccupante. Chiudo, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche ribadendo il ringraziamento, Presidente, nei confronti del ministro Lollobrigida, del ministro Schillaci e - attraverso lei - anche nei confronti della collega Maiorino.

in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali». *(Segue la

e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.200 (già

aumenta da 10 a 20 milioni, per gli anni dal 2023 al 2031, i fondi per monitorare gli ambienti chiusi sulla presenza del radon. Parliamo di scuole, di asili e anche di atenei e uffici.

Perché - ci chiediamo - non attingere i fondi dalle cosiddette riserve speciali? Capisco sia un impegno finanziario pesante, ma qui si tratta di prevenzione nell'ambito

il grande patrimonio biologico della nostra Nazione. Pertanto, questo emendamento

contiene una serie di norme particolarmente importanti che intervengono sull'annosa e complessa vicenda dell'ex Ilva, della quale ci siamo occupati non più di quattro mesi fa. Devo dire che ci aspettavamo che il Governo presentasse un nuovo emendamento dopo il decreto di quattro mesi fa, ma non ci aspettavamo che questo avvenisse così presto avvenisse così presto e materializzando una serie di norme che oggi stiamo discutendo e che tra poco dovremo votare. Voglio mettere subito in evidenza che c'è un enorme problema di metodo, dal momento che non è possibile affrontare un tema così cruciale e per qualche verso drammatico come la vicenda dell'ex Ilva con un emendamento presentato all'ultimo momento dal Governo - dal ministro Fitto - con un tempo ridottissimo

reale coinvolgimento del Parlamento e, per esempio, della Commissione industria, che pure lungamente ha discusso di questo provvedimento qualche mese fa, e senza soprattutto alcun confronto con il territorio, con le istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, dell'impresa e con i cittadini. Vi è, però, soprattutto un enorme problema di merito, perché l'emendamento dimostra ancora una volta, da parte del Governo, una totale mancanza di visione e un'assenza totale di politica industriale per un comparto fondamentale come quello della siderurgia.

Devo ammettere, signor Presidente, che è sempre sgradevole citare sé stessi e io di solito non amo farlo. In questo caso, però, non posso esimermi,

di fronte a una situazione debitoria pregressa e però c'era il rischio di bruciarne ancora, per via di una gestione che ogni giorno appare più discutibile e inadeguata. Il decreto-legge di qualche mese fa - ricordo la discussione che ci fu in quest'Aula - avrebbe dovuto rappresentare per il Governo una svolta, la possibilità di una continuità aziendale. alla luce di quello che stiamo vedendo e anche delle norme che oggi vengono presentate, la situazione è più grave di quella di quattro mesi fa: gli investimenti non ci sono stati e le scelte di allora oggi si sono rivelate un autentico fallimento. Noi allora avevamo proposto un percorso del tutto diverso, una soluzione alternativa e credibile rispetto allo scenario che si era venuto a creare. Avevamo chiesto di presentare un accordo di programma anche per dare un riconoscimento pubblico legislativo alla sofferenza della vicenda che ha riguardato Taranto nel corso di questi anni. Ma quell'accordo di programma, che pure era stato evocato dal ministro Urso, è rimasto lettera morta. Avevamo chiesto un piano di investimenti che però non c'è stato, anzi si continua a ricorrere alla cassa integrazione. Avevamo chiesto di realizzare una nuova *governance,*

perché elettrificazione e decarbonizzazione sono le strade che possono consentire a Taranto di ritornare centrale in Europa nella produzione di acciaio *green.* Oggi, con le norme che sono con le norme che sono state presentate, c'è il rischio di tornare indietro rispetto a tutto questo e di non affrontare quegli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di formazione dei lavoratori ai nuovi processi produttivi che sarebbe stato necessario fare. Non solo. Allora avevamo chiesto di limitare lo scudo penale, anzi di evitarlo o almeno di limitare la sua ampiezza ai fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute. Con questi emendamenti quello scudo penale viene ampliato e viene reso possibile anche per le opere del piano

locali, e che si configurano per quelle che sono, e cioè un accordo del Governo, forse un accordo del ministro Fitto con ArcelorMittal,

assegnato alla società di gestione, e cioè a quel socio privato che tanto l'ha osteggiato. Sarebbe anche importante che il ministro Fitto prima o poi ci dicesse che cosa sarà del PNRR e se le risorse legate al piano di decarbonizzazione verranno spostate al fondo di coesione, perché, se così fosse, ci vorranno anni in più, almeno due, se le cose dovessero andare bene. Concludo dicendo che noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che va ancora una volta nella direzione di correggere quello che il Governo ha proposto, perché vorremmo evitare che tutto questo si concludesse in un'ennesima occasione mancata, con il rischio di dover ritornare sulla

Paolo Borsellino cessava di vivere. Paolo Borsellino, un grande eroe italiano, un uomo che ha dedicato la propria vita al bene della comunità nazionale, affrontando a testa alta la criminalità organizzata, senza mai tirarsi indietro, senza mai cercare ribalte mediatiche. Il suo insegnamento è patrimonio comune e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della legalità e della giustizia. Quel 19 luglio del 1992, insieme a Paolo Borsellino, persero la vita anche gli agenti della scorta, servitori dello Stato: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, che è anche la prima donna della Polizia a perdere la vita in servizio. Personalmente, per i valori che hanno sempre ispirato il mio impegno in politica e anche per il mio particolare attaccamento alla Sicilia, vivo quel 19 luglio come una profonda ferita, che non si rimargina. Ma sono certo che non è solo mio questo sentimento, sentimento per un vile attacco al cuore dello Stato, di fronte al quale il nostro Paese seppe però trovare la forza di reagire con orgoglio, coraggio e dignità. Sono tanti i giovani che, da quel 19 luglio, da quella rabbia, da quell'indignazione, si sono avvicinati all'impegno civico per sconfiggere la criminalità in tutti i campi. Si rafforzò la convinzione che le mafie sono un cancro da combattere con determinazione, senza sconti, giorno dopo giorno. Le idee di Paolo Borsellino devono andare avanti con il nostro impegno, con le gambe delle nuove generazioni. Quella di Paolo Borsellino è un'eredità pesante, ma importante,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 Oggi con le nostre coscienze, con il cuore, con tutte le nostre storie di vita e di politica, pur diverse, sono certo, certissimo, che ci sentiamo tutti idealmente in questo momento presenti in via D'Amelio a onorare Paolo Borsellino. Sono esattamente trascorsi da pochi secondi i tempi, il minuto esatto in cui scoppiò quella tragica bomba, ed è in concomitanza di questo momento che vi prego di rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio per Paolo Borsellino e per tutti i caduti di mafia.

intervengo in merito a una serie di emendamenti che abbiamo presentato per cercare di correggere quanto proposto dal Governo: mi riferisco prettamente al tema e alla questione dell'Ilva. Il Governo aveva già introdotto una serie di norme come lo scudo penale e un finanziamento di 680 milioni di euro senza pretendere garanzie, assicurando una continuità senza introdurre delle tutele ambientali e sanitarie. In questo provvedimento, però, signor Presidente, il Governo si è veramente superato superato per una serie di ragioni, innanzitutto calpestando la Costituzione e dimenticando che ci sono due diritti costituzionali, il diritto alla salute e il diritto dell'ambiente, che vengono completamente schiacciati dal provvedimento nella sua interezza, calpestando altresì la dignità di un territorio che è stato considerato dall'ONU un territorio di sacrificio.

attivando tutti gli altiforni e senza introdurre alcuna tutela ambientale e sanitaria. Il Governo si supera tuttavia anche nell'ambito della reintroduzione dello scudo penale, perché va oltre quello che aveva già introdotto in termini di scudo penale sugli amministratori a marzo, ed estende lo scudo penale anche al dopo decarbonizzazione. Questa è una vera e propria assurdità: è come se la decarbonizzazione non servisse a nulla, dato che si introduce poi lo scudo penale anche per il periodo post-decarbonizzazione.

quindi, il diritto a uccidere, sia per lo scudo penale, sia per la possibilità di proseguire la produzione anche quando termineranno i tre gradi di giudizio e ci sarà

saranno i tempi della decarbonizzazione, perché nel PNRR il territorio aveva la certezza che entro il 2026 la decarbonizzazione doveva realizzarsi. Oggi, con questo provvedimento, abbiamo una doppia incertezza: non abbiamo più le risorse a disposizione (1,2 miliardi) e non abbiamo più i tempi della decarbonizzazione.

Vi è poi il tema della giustizia, quello di aver depotenziato anche la magistratura. Vorremmo denunciarlo, perché

una fabbrica che produce morte e malattia. Quindi, anche il conflitto di poteri tra Esecutivo e magistratura viene acuito con questo provvedimento, dando la possibilità allo stesso Presidente del Consiglio di andare a impugnare una sentenza

fuoco. Con questo emendamento chiedo che venga posta attenzione alla situazione, in particolare delle isole minori della Sicilia, perché una quota di questo organico che verrà impiegato, assunto a tempo indeterminato, possa essere riservato alle isole minori della Sicilia che attualmente non dispongono di un presidio continuo sul territorio. Sto parlando di isole che si trovano anche a due ore e mezzo di navigazione

la possibilità di rivolgersi a un presidio sul territorio. Tenuto conto che i periodi dell'anno in cui il presidio non è presente sono proprio quelli in cui le condizioni metereologiche sono particolarmente avverse, è facile immaginare in che situazione si potrebbero trovare gli abitanti dell'isola, quando per esempio vengono sospese le navigazioni per le condizioni del mare. Vorrei quindi invitare il Governo e la maggioranza a valutare l'opportunità di riservare una quota del numero di Vigili del fuoco che verranno integrati per le isole minori della Sicilia.

l'emendamento 18.204 interviene su una modifica approvata in Commissione che introduce all'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione il nuovo comma 1-*bis*, che dispone come contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata per gli stranieri che si presentino sprovvisti dei requisiti per l'ingresso sia ammesso il ricorso al TAR. L'emendamento riporta la giurisdizione sui restringimenti al giudice ordinario, come d'altronde è già oggi, perché così ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2014. La scelta del Governo verso il giudice amministrativo, che è il giudice della violazione degli interessi legittimi, invece che al giudice ordinario della sezione peraltro specializzata in materia di immigrazione del tribunale, non è corretta. Il respingimento può infatti avvenire anche nei confronti dello straniero titolare di diritti soggettivi di ingresso, quali: libertà di circolazione e soggiorno per i familiari extra Unione europea di cittadini dell'Unione, diritto di asilo, diritto di salute (per esempio, visti d'ingresso per cure mediche), diritto all'unità familiare.

riguarda il settore della vendita diretta a domicilio, che in Italia costituisce un comparto in continua espansione, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante all'interno del tessuto economico e occupazionale italiano, con un fatturato nel 2021 di 2,64 miliardi di euro, per circa 700.000 incaricati. La direttiva n. 2161 del 2019 sulla protezione dei consumatori ha prolungato da a trenta giorni il diritto di recesso solo per i contratti conclusi durante visite a domicilio non richieste, attraverso pratiche commerciali o di vendita aggressiva o ingannevoli. Nel gennaio 2023, il decreto legislativo n. 206 del 2005 ha recepito nell'ordinamento italiano la citata direttiva e conseguentemente ha aggiornato il codice del consumo. in fase di recepimento, il legislatore ha scelto di prolungare a trenta giorni il termine di recesso per tutti i contratti stipulati, nel contesto di visite a domicilio non richieste, senza alcuna distinzione rispetto alle modalità con cui questi sono svolti. una scelta che va in senso contrario, quindi, sia al dettato europeo in materia, sia alle richieste unitarie di tutto il settore. La proposta in esame, quindi, allinea le disposizioni nazionali a quelle europee, richiamando più chiaramente gli articoli del codice del consumo in materia di vendite aggressive e ingannevoli. Questo è un emendamento proposto dalla maggioranza. è piaciuto e non abbiamo compreso perché non lo si voglia più votare da parte della maggioranza, visto che amplia i diritti dei consumatori.

e da una contrattazione sfavorevole al primo produttore agricolo, che vede spesso, anzi quasi sempre, purtroppo, i prezzi di vendita non riuscire a coprire nemmeno i costi di produzione. Ne parliamo sempre, ma è necessario vedere l'interesse e l'intenzione del Governo a risolvere in qualche maniera delle problematiche ormai da tutti riconosciute. In questo ordine del giorno si puntualizza quali sono quali sono gli interventi auspicabili, come un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli alle piattaforme commerciali, favorendo gli accordi con la grande distribuzione, necessari per far sì che il prezzo possa essere equo per tutta la filiera. Quindi, parlare di filiere significa parlare anche del loro controllo, affinché affinché il prezzo e gli utili siano distribuiti in maniera equa su tutta la filiera. Altrimenti la produzione va a discapito della qualità, della sostenibilità ambientale e anche della copertura e

alla mercé del mercato internazionale, che non vede garantiti i costi, anche per la manodopera differente e i costi di gestione, che in Italia sono superiori rispetto all'estero. inoltre favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla prossimità territoriale, per evitare costi inutili di trasporto, anche per rispetto dell'ambiente. Il mio è un suggerimento al Governo, che spero voglia accogliere questo ordine del giorno, per dare un segnale importante al settore

Signor Presidente, desidero, a nome di Fratelli d'Italia, associarmi con ogni calore a questa grande notizia, questa grande notizia, che è arrivata - come ha detto il senatore Sensi - grazie all'impegno, soprattutto, di tantissime persone, organizzazioni non governative, associazioni, opinione pubblica, che sono quelle che hanno poi sostenuto, da sempre, anche la conclusione, purtroppo vicenda che ha riguardato il nostro connazionale mai dimenticato, neanche per un secondo, Giulio Regeni. Vorrei, in particolare, rivolgere un segnale di forte, attento e doveroso riconoscimento all'azione svolta dal Governo italiano, dal Governo del presidente Meloni,

si sgombra un'enorme nuvola nei rapporti fra Italia ed Egitto. Ed è veramente con grande soddisfazione che il Gruppo Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di un passo da parte egiziana così decisivo, ma così condiviso, senza clamori, senza battere pugni sul tavolo, senza alzare troppo le voci, ma facendosi valere in modo serio e determinato

tutta l'Italia è stata in pena e in pensiero per Patrick Zaki, un ragazzo egiziano che correva dei rischi serissimi nel suo Paese; certamente un ragazzo che abbiamo tutti in qualche modo adottato, le cui sorti non erano più soltanto un puro fatto di politica interna nel quale non ci si poteva intromettere. Era sicuramente interesse dell'Italia, volontà dell'Italia che fosse restituito alla sua vita, alla sua famiglia, alle persone che gli vogliono bene e anche alla sua Università di Bologna. Voglio riconoscere anch'io il lavoro del Governo e soprattutto il lavoro della Farnesina, il lavoro dei diplomatici della Farnesina che sempre, qualunque sia il Governo, di destra o sinistra, si distinguono sempre per essere tra i migliori del mondo. Voglio ringraziare personalmente l'ambasciatore Quaroni e tutto il suo *team* al Cairo, che hanno seguito il caso. Voglio dire, però, che certamente questa soluzione positiva migliora e alleggerisce i rapporti tra Italia e l'Egitto, che sono stati colpiti - diciamocelo chiaramente - dalla sentenza improvvisa di ieri, uno schiaffo in faccia al nostro Paese.

il presidente al-Sisi e l'ambasciata egiziana qui a Roma che questo esito positivo, del quale ovviamente ci compiacciamo, abbia risolto anche l'altra questione, perché la necessità di giustizia per Giulio Regeni è importante. È importante che finalmente gli atti della procura di Roma siano recapitati a chi li deve ricevere e che il percorso della giustizia non si fermi.

Signor Presidente, anch'io, a nome del mio Gruppo, esprimo la felicità per questa notizia. Abbiamo seguito, nella scorsa legislatura, come Commissione per i diritti umani, il caso di Patrick Zaki; abbiamo avuto modo di parlare anche con il nostro ambasciatore in Egitto e abbiamo cercato di essere di aiuto nella gestione di questa difficile vicenda,

un Paese che poteva sentirsi per questo messo sotto attacco. Oggi, quindi, si conclude questo percorso, anche se effettivamente di situazioni come quelle di Zaki ve ne sono

Presidente, anche a nome del MoVimento 5 Stelle mi unisco alle felicitazioni per

di fino, come ha detto il presidente Terzi di Sant'Agata. *(Applausi)*. Penso anche alla Commissione per i diritti umani, alla nostra senatrice Montevecchi, che aveva veramente portato avanti e sostenuto la causa

svolto in silenzio ma con efficacia - perché in casi del genere non aiuta il clamore della stampa - è riuscita in questo risultato. Vorrei anche rivendicare l'azione della Commissione esteri e difesa del Senato, che è andata in missione in Egitto qualche mese fa.

Provo ad aggiungere una riflessione. Molto spesso noi occidentali dimentichiamo che per quei Paesi i diritti umani significano accesso all'acqua, alle cure e all'alimentazione

come quello svolto con grande intelligenza dalla nostra diplomazia, riusciremmo a ottenere il rispetto dei diritti umani che chiediamo.

portata avanti e che deve continuare, perché non bisogna mai dimenticare che quello stesso Governo e quello stesso Presidente non ci hanno dato la possibilità di dare una giusta

altresì un grande ringraziamento alla diplomazia italiana, che ancora una volta ha dato una grande prova di sé nella capacità di tessere i rapporti, di mantenere salda l'attenzione e la concentrazione, fino ad arrivare a un risultato tanto atteso quanto a a volte anche insperato, proprio perché le condizioni della detenzione avevano fatto temere il peggio e poi invece ci sono stati, per fortuna, gli arresti domiciliari fino al provvedimento finale.

tuttavia non osservare, anche facendo seguito all'intervento della senatrice Craxi, che i Paesi del Nord Africa sono la nostra naturale controparte, sono dei *partner* commerciali importanti, sono strategicamente rilevanti sull'asse del Mediterraneo. Con loro dobbiamo cercare sempre di più di di ragionare e discutere di diritti umani, ma anche di politiche commerciali, di strategie sui flussi migratori e quindi lavorare sinergicamente con loro per lo sviluppo del Mediterraneo, nel rispetto dei diritti di tutti.

Signor Presidente, naturalmente in attesa della ufficializzazione di quanto ci è stato comunicato tramite agenzie e dei commenti che spettano innanzitutto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, non posso che aggiungermi ai sentimenti di di felicità, di sollievo e di compiacimento che sono stati espressi nell'Aula del Senato da tutti i Gruppi parlamentari.

del Governo, ma in realtà anche degli Esecutivi precedenti, di tutti coloro che hanno lavorato per la soluzione di questo caso umanitario.

Se sarà confermato, come speriamo, questo è un grande successo del Governo, ma in realtà dell'Italia e del Paese intero. Auspicando ancora una volta che questa notizia possa essere presto ufficializzata e confermata anche attraverso i canali

La Presidenza si associa ai sentimenti di soddisfazione espressi da tutti i Gruppi, augurandosi che le vicende abbiano il più concreto e rapido epilogo nel senso delle notizie che ci sono pervenute. La Presidenza esprime anche apprezzamento per l'azione che certamente sia i Governi precedenti che l'attuale Governo, con il presidente Meloni e il vice presidente Tajani, hanno svolto per assicurare un tale risultato.

vorrei invitare i colleghi a leggere questo emendamento, che abbiamo già discusso ampiamente in Commissione.

che sono classificate come zona scolastica e zona residenziale urbana, come previsto dal codice della strada, nonché su quelle aree nelle quali sono presenti ospedali e attività sanitarie in genere. Pertanto, rispetto ai due precedenti che avevano un impatto più ampio, specialmente in quelle viabilità cosiddette di scorrimento (quelle previste dal codice della strada a 70 chilometri orari), questo emendamento emendamento fa venir meno anche le osservazioni portate dal Governo e dalla Sottosegretaria per appoggiare o avvalorare la contrarietà. Invito i rappresentanti del Governo a valutare con attenzione questo emendamento, solo per la parte della lettera *b*-bis), perché stiamo parlando di ridurre non solo la velocità,

nello specifico di qualità dell'aria in prossimità di scuole, ospedali e edifici di culto, dove ci sono

l'emendamento 9.202, o proporre eventuali riformulazioni che possano rendere accoglibile la nostra proposta.

i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione del decreto legge convertito con la presente legge,

5a Commissione comunica che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201,

l'ottimo rischia di essere nemico del bene. Pertanto, per salvaguardare la riformulazione che prima veniva citata e che - lo ricordo - è stata approvata all'unanimità da parte di tutti i Gruppi, noi ritiriamo la richiesta che a nostro avviso andava fatta - poi lo spiegherò in dichiarazione di voto - e cioè di anticipare al 2023 e al 2024 il risultato buono che noi abbiamo raggiunto nella riformulazione.

Procedo con ordine. È vero che tutti i Gruppi hanno presentato emendamenti su questa materia, che è il tentativo di provare a mettere ordine al personale precario Alta formazione che non tutti i Gruppi hanno seguito le stesse indicazioni, né hanno raccontato le stesse soluzioni delle vicende che vive il personale Afam. Noi siamo stati contenti, quando il Governo ha proposto una riformulazione, partendo dagli emendamenti del senatore Lombardo, che però comprendevano anche il testo presentato dal Partito Democratico a prima firma del

che abbiamo considerato accettabile, a patto che - e questo il Presidente relatore lo sa - il relatore si impegnasse in un ulteriore emendamento, che poteva trovare l'accordo di tutte le forze politiche, che è quello nella versione degli

che sono diversi dagli accordi che erano stati fatti. Allora, io penso che al netto di tutto - e apprezzo le parole del collega Lombardo, che vuole portare a casa il risultato, e lo comprendo, perché nel testo il risultato c'è

dà un incremento di dotazione al personale dei Vigili del fuoco. Ora, io penso che questo tema sia caro a tutti; c'è un'infrazione in corso anche su questo. Il Governo in questa direzione avrebbe dovuto fare

Signor Presidente, vorrei solo ricordare che, con il voto contrario a questo emendamento, state dicendo "no" ai cittadini delle isole minori della Sicilia a un presidio permanente sulle loro isole, che per questioni di logistica sono nettamente svantaggiate in caso di emergenza. Non essendoci un presidio costante sull'isola, quella popolazione la abbandoniamo a se stessa. Quindi, prendetevi le responsabilità di questo voto contrario.

**Il Senato non approva**.

che la ricostruzione della carriera del personale della scuola avverrà secondo regole che vanno a toccare i diritti acquisiti, perché si cambia completamente il calcolo. è stato considerato quale sarà il costo di tutti i ricorsi che verranno fatti, ma di questo parleremo. L'emendamento in realtà chiede che anche le scuole paritarie - non sono le scuole pareggiate, perché il termine "pareggiate"

delle scuole paritarie o che hanno prestato servizio anche nelle scuole paritarie gli stessi diritti riconosciuti agli altri insegnanti Se la maggioranza vota contro questo emendamento, che modifica una dicitura che - lo ripeto - non c'è più, perché le scuole pareggiate sono un'altra cosa dal 2000 in avanti,

Posso dire infatti che, quando siamo stati capaci di lavorare insieme, anche nelle leggi di bilancio, abbiamo costruito proposte emendative comuni e trasversali. Mi chiedo dunque per quale motivo non ci sia ora la volontà di modificare questo termine, inserendo tutte le scuole certificate all'interno del sistema nazionale di istruzione; diversamente, rischiamo altri ricorsi, ma, soprattutto, una classificazione

all'interno di questo provvedimento si cerca di sanare un'ulteriore infrazione in cui è incorsa l'Italia. È l'infrazione che riguarda il *bonus* docente che era stato attribuito solo al personale di ruolo e non al personale precario. Che cosa ha detto l'Europa? Attenzione: noi dobbiamo riconoscere tutti gli insegnanti esattamente allo stesso modo. Questa - ve lo dico - era una riflessione che era nata anche quando abbiamo approvato la legge n. 107 del 2015, cosiddetta buona scuola, senza che ce lo dicesse nessuno. avevamo istituito questa norma, la cosiddetta carta docente, che garantisce 500 euro ad ogni docente per l'autoformazione. Avevamo detto di partire dal personale di ruolo, anche perché - prevengo qualsiasi critica siamo stati gli unici che hanno assunto personale di ruolo docente per 100.000 unità: il più grande piano di assunzione. Oggi l'Europa ci dice che è necessario che i 500 euro vengano dati anche al personale precario. Cosa fa il Governo? Non considera tutto il personale precario, ma considera quello che è sulle cattedre libere dal 1° settembre al 31 agosto, non considerando invece tutti i docenti che fanno supplenza anche dal 1° settembre al 30 giugno, e sono tante cattedre e tanti lavori che potremmo considerare completi e per tutto l'anno scolastico. Allora, penso che la maggioranza anche qui, onde evitare nuovi ricorsi e nuovi contenziosi e quindi di dover far pagare il Paese, dovrebbe appoggiare questo emendamento e votare a favore.

noi abbiamo espresso sugli emendamenti 11.202 e 11.203 parere non ostativo condizionato, *ex* articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione emendamenti 11.200 e 11.201, ma la riformulazione si accetta in Aula, perché la nostra Commissione dà solo pareri finanziari. Quindi, non è corretto dire 5a Commissione ha consentito la riformulazione degli emendamenti, perché le ricordo che noi siamo in sede consultiva e non referente. Quindi, non possiamo toccare nulla in quella Commissione. anche rispetto ai colleghi, altrimenti si rischia di dire cose che poi non sono vere nella realtà.

intervenuta. Si è riaperta una discussione sull'articolo 11. Se vuole può parlare un minuto, ma comprenda che è un po' irrituale sia parlare dell'articolo 11, sia che lei riprenda la parola.

qualora fossero stati riformulati in quel modo. Sono due emendamenti completamente diversi. Lei può dirmi "non lavoriamo nel merito", ma non era accettabile questo tipo di interpretazione qui in Aula non da lei, ma da chi avrebbe dovuto dirci come mai non ha presentato l'emendamento in quanto relatore.

Presidente, sull'emendamento Scurria, trasformato in ordine del giorno, il Governo dà un parere favorevole, previa riformulazione Governo: a valutare l'opportunità di prevedere forme sempre più avanzate di tutela dei consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli,

l'abbiamo fatto nostro, dopo che la maggioranza non lo ha ritirato, avendo avuto il parere contrario. Non riesco a capire come questo emendamento possa essere diventato un ordine del giorno del senatore Scurria e, quindi, mi rifaccio eventualmente a meccanismi che mi sfuggono e chiedo scusa. Non riesco però a capire come mai questo sia diventato un ordine del giorno di un senatore che quell'emendamento - mi spiace dirlo - non l'aveva più, perché

della Commissione, perché l'Assemblea fa il suo esame. C'è stato un parere, il Governo ha anche condizionato il parere favorevole a una riformulazione che il presentatore ha accettato. Quindi, in termini parlamentari è una procedura assolutamente corretta; poi l'Assemblea decide. Malpezzi, ha parlato tutte le volte che lo ha chiesto e anche di più.

un ordine del giorno presentato al posto di un emendamento. Abbiamo semplicemente un ordine del giorno che viene presentato in Aula. Il punto politico che stava segnalando la senatrice Malpezzi è che il proponente dell'emendamento voterà probabilmente contro il suo stesso emendamento. Questo è semplicemente un punto politico, perché era un suo emendamento che è stato presentato nel testo. È solo per dare chiarezza rispetto a quello che è avvenuto in Commissione. lei dovrebbe avere imparato che l'ordine del giorno è cosa diversa da un emendamento, perché è un auspicio, la cui formula è: «impegna il Governo a valutare l'opportunità»; poi, il Governo ha posto delle condizioni.

A questo punto, per far capire all'Assemblea e a ciascuno di noi cosa stiamo facendo, essendo state accettate queste riformulazioni, abbiamo dei testi identici.

ma in realtà è uno strumento normativo estremamente utile per l'Italia. Parliamo del decreto-legge salva infrazioni che - come si evince dal nome stesso - ha l'obiettivo di scongiurare o quantomeno ridurre le procedure di infrazione già avviate da parte dell'Unione europea nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovi procedimenti rispetto a quelli già esistenti. Ringrazio il Ministro e il Governo che hanno proposto questo provvedimento che abbiamo esaminato in Commissione nelle ultime settimane.

Le procedure sulle quali si interviene afferiscono a diverse materie. Per questioni di brevità non spetta al sottoscritto citarle tutte, ma vorrei evidenziarne solo alcune: dalle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, per cui varrà il criterio non più di cittadinanza, ma di residenza, alla disciplina del personale volontario a tempo determinato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle disposizioni che riguardano le modifiche al codice della strada. In questa fattispecie, fra l'altro, si prevede che Regioni e Province autonome, sentiti i prefetti, possano disporre la riduzione della velocità nelle strade extraurbane, nei tratti che attraversano centri abitati o in prossimità

Siamo di fronte a una rivoluzione culturale. Come ha pubblicamente detto il ministro Pichetto Fratin, si modifica il codice della strada non solo per motivi di sicurezza stradale, ma anche - come in questo caso - per ragioni legate alla tutela dell'ambiente. Un altro dispositivo normativo sempre in materia di ambiente è quello che prevede divieti sugli abbruciamenti dei residui agricoli proprio per limitarne l'impatto sulla qualità dell'aria.

Cambiando completamente settore, alcune disposizioni previste dagli articoli 11, 14 e 15 riguardano rispettivamente il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni AFAM, il riconoscimento per il personale docente e amministrativo,

dei docenti di ruolo, per un importo di 500 euro a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile. Sono norme che rappresentano un passo in avanti nella giusta direzione, una prima risposta importante per il personale del comparto della scuola, in ottemperanza alle disposizioni europee. con un passaggio sullo sport. Siamo ben consapevoli di quanto l'attività sportiva svolga un ruolo chiave nelle nostre comunità come strumento di crescita oltre che di promozione del benessere e di uno stile di vita sano.

a condizione che gli stessi utili siano destinati allo sviluppo di attività statutarie non commerciali. Credo sia un passo in avanti importante, anche perché - come ha detto il ministro per lo sport e i giovani Abodi - lo sport è la difesa immunitaria sociale delle nostre comunità

preventivo con la Commissione, che evita l'apertura di procedure di infrazione. Per queste ragioni, come Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-MAIE, annunciamo il nostro voto favorevole. Presidente, Governo, colleghi, credo che oggi stiamo perdendo l'ennesima occasione per sanare alcune criticità, seppure vi siano degli elementi positivi che, come Alleanza Verdi e Sinistra, non disconosciamo. Per esempio, l'articolo 11 tratta delle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (procedura di infrazione n. 2014/4231). Si tratta di una norma particolarmente attesa, in quanto prevede il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo sia del personale amministrativo che del personale docente. Con tali modifiche, a decorrere dal 14 giugno 2023, a tutto il personale che abbia svolto servizio a tempo determinato o in un ruolo inferiore per più di quattro anni tale servizio deve essere valutato per intero e non per i due terzi, per la parte eccedente i quattro anni. Naturalmente il provvedimento non riguarda eventuali arretrati degli anni precedenti, per i quali la strada rimane quella del contenzioso. Inoltre, è disposta l'estensione dell'imposta di registro agevolata prima casa per l'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o lavorava prima del trasferimento. Novità, inoltre, ci sono anche nel settore dello sport. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. Tuttavia, risulta non ancora centrato il diritto di veder riconosciuta, al personale degli enti di ricerca, l'anzianità di servizio pre-ruolo svolta anche con contratti atipici. Pertanto, sarebbe stato opportuno modificare il provvedimento, senza alterare la finanza pubblica, prima della legge di bilancio, impegnandosi subito per le stabilizzazioni. Avevamo chiesto, come altri Gruppi, di prevenire il probabile avvio di ulteriori procedure di infrazione attraverso la progressiva stabilizzazione del personale precario con almeno tre anni di servizio, tenendo altresì conto - da un lato - delle modifiche in tema di reclutamento previste dall'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale e - dall'altro - delle notevoli responsabilità organizzative attribuite alle singole istituzioni AFAM. Abbiamo chiesto che la carta di 500 euro l'anno prevista per l'aggiornamento dei docenti fosse concessa anche al personale docente a tempo, non distinguendo tra docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (termine del 31 agosto) e docenti con supplenza annuale su posto non vacante, ma di fatto disponibile Si tratta di oltre 130.000 posti, la maggior parte dei quali attiene ai contratti conferiti su posti dati in deroga sul sostegno, che sono in continuo aumento. Pertanto, al fine di evitare ulteriori discriminazioni e conseguenti contenziosi, crediamo sia necessario estendere il beneficio della carta elettronica a tutto il personale docente con supplenza annuale, sia esso su posto vacante, sia esso su posto non vacante, ma disponibile fino al termine delle attività didattiche. insegnanti sono gli eroi del nostro tempo e non è giusto continuare a non valorizzarli. Non ultimo, abbiamo chiesto che la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del sito dell'Ilva di Taranto di Taranto rimanessero in seno al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (non più della transizione ecologica) e non alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di valutazione ambientale andrebbero definiti dal Ministero dell'ambiente e andrebbe rafforzato il finanziamento economico del processo di decarbonizzazione, che resta fermo al limite di 150 milioni di euro. L'assenza ancora una volta di risposte certe, con la previsione di risorse e l'adeguamento dei fabbisogni per realizzare le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, non può che vederci in totale disaccordo. Pertanto annuncio il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento Signor Presidente, ci troviamo ormai in pochi a discutere la conversione in legge di un decreto decreto importante sotto vari profili e sotto diversi punti di vista. Perdonatemi se, prima di entrare nel merito del provvedimento, farò un preambolo sul metodo. metodo. Non solo purtroppo ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge e all'ennesima decretazione d'urgenza che comprime le prerogative di quest'Aula e della funzione dei parlamentari, ma lo strumento principale perché l'Italia si adegui agli obblighi derivanti dall'Unione europea esiste ed è la legge, Pertanto, come ribadito dal presidente della 4a Commissione Terzi Di Sant'Agata, mi auguro che il Governo si prenderà l'impegno di adottare la legge europea e la legge di delegazione europea, evitando la decretazione d'urgenza quando bisogna adeguarsi a degli obblighi europei. Andiamo adesso nel merito del provvedimento, un provvedimento corposo che riguarda 38 articoli, di più dei 27 originali. Ci sono diverse cose positive, altre meno. Innanzitutto con questo provvedimento noi chiudiamo diverse procedure di infrazione e di pre-infrazione e ci adeguiamo anche a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, riportando l'Italia

il collega, senatore Filippo Sensi, quando in Commissione ha detto che è un provvedimento lardellato di discrezionalità politica. Dico questo perché in Commissione più volte ho chiesto al ministro Pichetto Fratin e al ministro Fitto come mai sia stata scelta la chiusura di alcune procedure di infrazione e non di altre.

alla dichiarazione di doppia condanna segue il pagamento da parte dell'Italia di sanzioni pecuniarie per mancato adeguamento agli obblighi europei. poi nella parte delle conclusioni a come - a mio avviso - dovrebbe essere legata invece la fase discendente, che è quella della quale stiamo parlando, con la fase ascendente, ma lo dirò alla fine. cosa c'è dentro questo provvedimento? Ci sono tante cose. Ci sono temi come quello dell'Ilva, sul quale mi limito a dire che è la terza volta in nove mesi

Abbiamo votato a favore dei Vigili del fuoco e sarà difficile per la maggioranza spiegare perché il voto invece è stato contrario su un emendamento della senatrice Malpezzi. Abbiamo votato a favore di un emendamento dei giudici onorari, perché non è possibile che persone che svolgono la funzione giurisdizionale, pur non avendo vinto un concorso da magistrato ordinario, quindi col titolo di giudici onorari, non abbiano riconosciute le tutele in termini di maternità, di paternità e di profili pensionistici. Questa è una vergogna. Ma vorrei concentrare l'attenzione su due provvedimenti che mi stanno molto a cuore. Il primo riguarda il tabacco riscaldato: siamo soddisfatti che in sede di Commissione politiche europee del Senato sia stato sciolto il nodo relativo alla norma sul tabacco riscaldato per l'estensione del divieto di immissione sul mercato di prodotti con aromi caratterizzanti. bene recepire correttamente le indicazioni dell'Unione europea, ma perché è importante farlo per noi? Questo ha un notevole impatto per la manifattura e l'agricoltura italiana. Ricordiamo che nella filiera agroindustriale del tabacco riscaldato *made in Italy* lavorano 40.000 persone, per la realizzazione di prodotti altamente innovativi, con un forte radicamento su territori che conosco molto bene, perché questo stabilimento si trova a Valsamoggia e ho presenziato alla sua inaugurazione quando il Presidente del Consiglio era Matteo Renzi. C'è un'altra norma sulla quale voglio soffermare la mia attenzione e lo faccio rivolgendomi ai portavoce dei precari dell'alta formazione artistica e musicale che sono qui e ci stanno ascoltando, perché è un impegno che mi sono preso con loro e che ho cercato di portare avanti al massimo delle mie capacità. Qual è il tema, signor Presidente? L'Unione europea ci dice che non possiamo abusare di un contratto a tempo determinato, evitando la stabilizzazione di persone che lavorano nell'alta formazione artistica e musicale.

le senatrici della maggioranza che sono presenti qui in Aula, anche la senatrice Bucalo e tutte le persone che sono intervenute. Quando ho detto prima che a volte l'ottimo è nemico del buono, volevo dire

Era un errore sotto diversi punti di vista, perché non conteneva la valorizzazione di chi continua a lavorare in un precariato endemico e strutturale nell'alta formazione artistica e musicale. Noi a queste persone dovevamo dire che non solo l'Italia ha sbagliato nell'abusare del contratto a tempo determinato, ma è stata causa di quella precarizzazione endemica che oggi andiamo a risolvere. L'avremmo risolto in modo pieno se avessimo anticipato tutto questo al 2023. Tuttavia, piuttosto che tornare indietro rispetto al testo che all'unanimità, nel riconoscimento delle prerogative della funzione parlamentare, abbiamo ottenuto, mi sono sentito, in accordo con il presidente Terzi di Sant'Agata, di ritirare il mio emendamento, perché la parola data ha un un valore nel momento in cui la nostra priorità doveva essere salvaguardare quel testo 2 che è merito di tutti se abbiamo approvato in Commissione. Qual è il nodo, Presidente, rispetto a questo tema? Che cosa manca? Manca il regolamento per l'abilitazione nazionale: è questo che manca. l'idea di prevedere un concorso riservato per chi ha svolto queste attività non è solo un messaggio di fiducia nella politica e nelle istituzioni, e di dignità del lavoro svolto, ma ha anche un altro significato che per me è molto importante: riconoscere che chi lavora nell'alta formazione musicale non è un semplice divulgatore di sapere e di conoscenza, bensì un creatore di sapere e di conoscenza *(Applausi)*, e come tale non deve essere attratto al sistema scuola, ma deve essere inserito nel sistema dell'università. È questo il punto che oggi noi affermiamo. Dobbiamo dire a tutte queste persone - sono tante, sono 1.700 che attendono questa risposta - che dovranno aspettare altri sei mesi; purtroppo non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo adesso. Credo però che, dopo un'attesa fatta di decine di anni, aspettare sei mesi in qualche modo sia un male minore. Presidente, annuncio a nome di Azione e Italia Viva il voto di astensione. Avremmo voluto votare favorevolmente. Ringrazio il Presidente per aver fatto svolgere alla Commissione politiche europee la sua vera attività. Se fosse stato dato l'ok e il parere conforme sul tema dei Vigili del fuoco, sul tema dell'anticipazione del 2023, sul tema dei giudici onorari, esprimerci in maniera positiva. Però - e con questo concludo - non è semplicemente lavorando sulla fase discendente degli obblighi dell'Unione europea che noi occorre lavorare nella fase ascendente. Voglio concludere con una citazione di un compianto sindaco di Bologna, che si chiamava Renzo Imbeni e che, se la politica italiana fosse stata più furba, l'avrebbe visto come Presidente del Parlamento europeo. Egli diceva che la sovranità nazionale si esercita consapevolmente nelle sedi europee e sovranazionali. Quando saremo arrivati ad assumere obblighi come direttive, regolamenti e decisioni, esercitando consapevolmente quella sovranità, allora probabilmente non avremo più bisogno di decreti salva infrazioni, perché vorrà dire che avremo imparato a difendere e a esercitare compiutamente quella sovranità a livello europeo.

posto che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero di procedure pendenti nei confronti del nostro Paese era di 83, di cui 39 per violazioni del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive. È per questa ragione che il Governo ha adottato lo strumento del decreto-legge: per diminuire questa lunga lista di inadempienze. Fino ad oggi ne sono state chiuse 11, mentre nel frattempo altre 10 si sono aggiunte a quelle precedenti. Ecco quindi che le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia oggi sono 82, mentre la media europea è di 66. Con il disegno di legge in esame è stato però possibile anche adottare provvedimenti necessari a fronte degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Quindi la finalità è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure, ovvero che si aggravino quelle esistenti. Di fronte alle 82 infrazioni aperte, il decreto-legge, dopo le opportune interlocuzioni del Governo con la Commissione europea, prevede di portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Oltre a ciò, è prevista l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea. Anche le misure introdotte in Commissione prevedono ulteriori interventi in materia di adempimento di obblighi europei. Come ha detto ieri il nostro Presidente e anche relatore Terzi di Sant'Agata, si arriva così complessivamente a 35 procedure risolte positivamente: questo porta l'Italia a raggiungere la media europea e a non trovarsi nella parte più negativa. Il decreto-legge in esame serve anche ad evitare possibili sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

Evitare nuove contenziosi e nuove sanzioni avrà quindi anche un impatto positivo sui conti pubblici, posto che comunque il nostro ordinamento è tenuto ad adeguarsi a quello comunitario. Questi dati così significativi ci consentono di sottolineare lo spirito autenticamente europeista di questo Governo, a fronte di chi invece alla vigilia paventava delle posizioni sovraniste che ci avrebbero posto in contrasto con gli organismi europei. Durante l'esame in Commissione sono state accolte alcune proposte del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE. Un emendamento riguarda le assunzioni straordinarie dell'AFAM, per cui, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono indire procedure di reclutamento straordinario. Un altro tema che abbiamo affrontato è quello della ricetta medico-veterinaria cartacea, che può affiancare quella elettronica in determinate circostanze. Il Governo ha recepito questa problematica, accogliendo un nostro ordine del giorno. Un altro punto accolto dal Governo è quello del tabacco riscaldato, per il quale sono state recepite alcune puntualizzazioni normative, relative a lavorazione, presentazione e vendita. Quest'ultimo è un importante intervento normativo, al fine di recepire in modo corretto un provvedimento comunitario particolarmente importante per la filiera del *made in Italy*, che punta alla sostenibilità delle produzioni e dei consumi. La norma va anche nella giusta direzione di non scoraggiare l'innovazione nel comparto, con produzioni che guardino anche a un minor impatto sulla salute pubblica. È una norma che il nostro Gruppo ha voluto e che ha visto l'accordo di tutta la maggioranza, insieme al Governo, ha lavorato con la Commissione, per definire la migliore formulazione possibile per trasporre quella direttiva delegata e per garantire una normativa nazionale chiara ed efficace, tenuto conto che l'Italia aveva espresso forti perplessità a Bruxelles sulla base delle definizioni di tale norma, anche relativamente al rispetto delle procedure decisionali unionali. Siamo soddisfatti di questa norma nazionale, che conferma l'attenzione di Forza Italia e della maggioranza all'allineamento agli obblighi comunitari, garantendo nel contempo la necessaria tutela del comparto produttivo nazionale e ponendo quindi una forte attenzione anche al corretto modo in cui recepiamo in Italia le norme che ci arrivano da Bruxelles. Complessivamente, nel decreto-legge sono state trattate molte altre tematiche. Mi permetto di soffermarmi da ultimo, *ratione materiae*, sull'articolo 18-*bis* in tema di mandato di arresto europeo, inserito per adeguare l'ordinamento interno alle più recenti interpretazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. disposizione interviene prevedendo la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza, anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano in Italia da almeno cinque anni. Ciò in quanto, secondo la Corte, è legittimo che lo Stato membro di esecuzione persegua il reinserimento sociale nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento. Signor Presidente, mi permetta, a conclusione del mio intervento, di ringraziare il presidente della Commissione Terzi di Sant'Agata, per il lavoro e il contributo, e anche il dottor Capuano e i collaboratori della 4a Commissione per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata, a supporto del nostro lavoro. Quindi confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE

almeno ai pochi colleghi rimasti in Aula ad ascoltare le dichiarazioni di voto. Signor Presidente, le chiedo un attimo di attenzione e approfitto della presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento, per mettere in evidenza ancora una volta

due leggi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Pertanto, anche grazie all'innovazione apportata alla fine del 2021,

a dover invece affrontare delle problematiche complesse, quali quelle legate alle procedure di infrazione in generale, con un decreto-legge che non ha neanche i requisiti dell'urgenza. Diciamo che ci sono dei precedenti, ma che risalgono alla XVII legislatura.

volte a dare un *assist* a questa scelta, che secondo noi non solo è inappropriata, ma continua a mortificare il Parlamento. il Parlamento. Nella scorsa legislatura c'era il collega Fazzolari, ora Sottosegretario alla Presidenza, che si alzava ogni qualvolta ne aveva l'opportunità, in Aula e in Commissione, additando gli allora Governi di turno perché comprimevano troppo troppo la discussione in Aula. Voi cosa state facendo? Avete utilizzato una via impropria, quando c'è già la possibilità. Pertanto, al di là di poter accettare, siamo a 10 mesi dall'inizio del nuovo Governo e ci auguriamo che, nel giro di breve tempo, il Governo ci porti la legge europea, all'interno della quale dovremmo andare ad affrontare temi ma con il Regolamento del Senato avremo la possibilità di farlo anche in maniera più snella. Ma è sicuro che, in questo modo, voi ci impedite di dare un contributo fattivo, perché è nell'interesse di tutti lavorare al meglio e trovare le migliori soluzioni possibili per evitare che le procedure di infrazione si trasformino in un peso economico per la Nazione.

Ricordo all'Aula - e i colleghi che seguono la questione lo sanno meglio di me - che vi è il precontenzioso, poi c'è la sentenza, ma solo dopo la seconda sentenza di condanna lo Stato membro deve sborsare per cento degli articoli riguarda un precontenzioso, mentre abbiamo tante altre procedure di infrazione, tra cui quella sui reflui industriali, dove invece abbiamo anche sentenze doppie, dove già paghiamo un un bel po' di soldi (circa 60 milioni di euro l'anno). Dobbiamo puntare l'attenzione più su quello che sui precontenziosi. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo già prevenire? Bene. Lavoriamo anche sulla prevenzione, ma facciamolo nelle sedi deputate e fate lavorare per bene i parlamentari perché noi siamo pagati per questo. Se mi permettete, passo a fare alcuni appunti su alcuni ordini al giorno che sono stati accolti in Commissione e di questo ringrazio sia il relatore che i colleghi ma anche i membri del Governo. Sono i temi che seguo dalla passata legislatura ed uno è legato all'incompatibilità tra professione dell'agente immobiliare e quella del mediatore creditizio. Noi eravamo riusciti, nella legge europea 2019-2020, che abbiamo chiuso nel 2021, a risolvere il problema legato all'infrazione. Solo che alla fine della scorsa legislatura, a Camere chiuse, sostanzialmente, con un colpo di mano è stata fatta una modifica che ha riaperto quella procedura. Ora con questo ordine del giorno, mi permetto, tramite il Presidente, di ricordare al ministro Ciriani e al Presidente della mia Commissione, di stare attenti, perché ora

all'ordinamento italiano che, in generale, dà la possibilità alle associazioni tra professionisti di fare una società finalizzata a massimizzare, a migliorare e rendere più efficace ed efficiente la propria azione. Per quanto riguarda

di quella fattispecie, perciò in generale quando si tratta di salute pubblica, sia messa al centro sempre la salute dei pazienti e per noi la via maestra è solo quella di creare società tra professionisti, perché gli odontoiatri sono anche tenuti a rispettare un codice deontologico.

Vi ringrazio per questo, ma il tema è trasversale. Penso che la salute sia un interesse e un obiettivo comune a tutti noi.

dei ricercatori e dei tecnici degli enti pubblici di ricerca. Anche in questo caso, poiché dobbiamo pensare a evitare la fuga dei cervelli, la loro ricostruzione di carriera è importante. Abbiamo su questo delle procedure di infrazione con le quali ci hanno bacchettato più volte, non ci possiamo permettere di tenere delle menti eccelse con contratti a termine rinnovati per decenni,

continua a bacchettare la popolazione di Taranto, perché non si risolve né il problema ambientale, né quello della salute. Costringiamo quei territori a dover scegliere se morire di fame o morire di cancro. morire di cancro. Non possiamo trattare in questo modo quei territori, siti di interesse nazionale per le bonifiche. Io vengo da Gela e quelle manifestazioni le ho vissute e le vivo sulla mia pelle. Parlare con i genitori di bambini malformati è una cosa terrificante. Non giochiamo con la salute della gente. *(Applausi)*. In conclusione, vi posso soltanto dire stare attenti. Il MoVimento 5 Stelle, proprio per questo emendamento, voterà contro il provvedimento, perché è ingiusto e immorale che si lucri sulla salute e sull'ambiente.

signor Ministro, l'Europa è un'organizzazione complessa, con un sistema legislativo molto articolato. Questo sistema è stato messo in atto per garantire che gli Stati membri seguano le stesse regole e norme, in modo da creare un mercato unico e garantire la tutela dei diritti dei cittadini europei. Mercato unico significa armonizzazione delle legislazioni nazionali per permettere alle nostre imprese di essere competitive sul mercato globale. Questo è il primo punto su cui lavorare per creare il vero mercato unico che è stato istituito nel 1993. Ad oggi, però, non funziona così. Dobbiamo farci concorrenza tra di noi nello stesso mercato europeo con un *dumping* fiscale e salariale. Questo sistema è diventato così complesso e ingombrante che sta diventando sempre più difficile per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione e inoltre sta portando a un aumento del numero di procedure di infrazione, che sono costose e dispendiose in termini di tempo per tutti gli interessati. Per risolvere questo problema è necessario semplificare il sistema legislativo dell'Europa, ridurre il numero di norme e regolamenti e rendere più semplice per gli Stati membri conformarsi al diritto dell'Unione. tendenza, invece, sembra andare in direzione contraria, soprattutto viste le nuove tematiche, come quella ambientale, o cosiddetta *green,* e la transizione industriale: ci sono decine di regolamenti che impongono specifici limiti, spesso inapplicabili, viste le peculiarità dei diversi Stati membri, e che porteranno ad un inesorabile aumento delle procedure di infrazione e a storture del mercato interno. Presenteremo un pacchetto di aiuti per le piccole e medie imprese, che comprenderà una proposta per un insieme unico di norme fiscali per fare affari in Europa, chiamato Befit e renderà più facile fare affari nella nostra Unione. Lo ha annunciato direttamente la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo del settembre 2022.

Ciò significa che non si tassano direttamente le imprese, ma gli Stati, tra cui l'Italia, dovranno dare un contributo in base al reddito che le stesse aziende avranno all'interno dell'anno fiscale. quindi oneri aggiuntivi in più per il nostro Paese. Gli oneri delle direttive europee, specialmente quelli del pacchetto Fit for 55, vanno a gravare sulle nostre aziende, specialmente le piccole e medie imprese che rappresentano il 99 per cento del tessuto imprenditoriale europeo.

con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi, che consentono di identificare l'odore e il gusto dei prodotti del tabacco interessati e la loro intensità di fumo.

Successivamente è stato approvato un emendamento sul servizio di interrompibilità del carico elettrico che, oltre ad accogliere le forti preoccupazioni del sistema industriale, si pone in linea con quanto espresso dalla Commissione europea, che ha chiesto di rivedere il meccanismo, anche prevedendo l'abrogazione delle norme in questione in occasione della naturale scadenza della procedura. Per quanto riguarda le quote latte, oggi abbiamo approvato direttamente in Aula un nuovo criterio di ricalcolo per il supplemento del latte per i soggetti destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione di prelievo supplementare e disposto il ricalcolo.

in materia di scuola, sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, al solo fine della partecipazione a procedure selettive, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se è stato svolto ininterrottamente dal 10 febbraio allo scrutinio finale. intervento, vorrei fare una sottolineatura e una precisazione. In Commissione abbiamo ritirato l'emendamento per il riconoscimento di carriera delle scuole paritarie perché necessita di una copertura. Questo Governo ha fatto tanto, anche nell'ultimo decreto PA2. Conosciamo il problema delle scuole paritarie e naturalmente di tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti devono essere uguali all'interno del sistema scolastico nazionale. Il problema naturalmente necessita di una copertura e quindi abbiamo valutato con il Governo di affrontare direttamente questa tematica nel prossimo provvedimento utile. Questi sono solo alcuni degli esempi di infrazioni corrette in questo decreto. Ma le battaglie nella Commissione politiche europee continuano ogni settimana, con pareri contrari motivati contro direttive europee insensate contro il nostro sistema nazionale. Il più evidente è stato quello che abbiamo approvato il 19 aprile, quando abbiamo inviato alla Commissione europea, sulla proposta di regolamento degli imballaggi, un parere naturalmente contrario con delle osservazioni, perché andava direttamente contro il sistema Italia, che è basato su un sistema di riciclo.

Di conseguenza possiamo concludere che l'Europa è un'istituzione che incarnava il sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei, ma si è trasformata negli anni in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare. Tali caratteristiche contribuiscono ad alimentare la diffidenza che i cittadini europei hanno verso le istituzioni comunitarie, viste come lontane dalla realtà e soprattutto inconciliabili con le differenti necessità e peculiarità degli Stati membri. È tempo di cambiare e i cittadini lo hanno capito, dando segnali forti nei Governi nazionali; lo faranno sicuramente anche alle prossime elezioni europee. Signor Presidente, signor Ministro, senatrici e senatori, il decreto-legge salva infrazioni, che discutiamo oggi, è una risposta sbagliata a una domanda sbagliata. sbagliata. Non lo dico - credetemi - perché sono all'opposizione e, per definizione e liturgia, si critica a prescindere qualsiasi provvedimento proposto dalla maggioranza. Ci sta, è il gioco delle parti, ne sa qualcosa il Gruppo Fratelli d'Italia: coerentemente all'opposizione nel corso della scorsa legislatura, opposizione facile, ma nitida, sulla quale Giorgia Meloni ha costruito tanta parte del suo successo elettorale e la sua lunga marcia verso Palazzo Chigi. Ne sa qualcosa però anche il suo *junior partner*, la Lega, - permettetemi questo punto politico - che ha pagato salatissimo, a mio modo di vedere, esattamente il contrario, cioè la mancanza di coerenza, l'appoggio intermittente a Governi di segno opposto e una linea di difficile comprensione per gli elettori. Infatti ha vinto Meloni e non Salvini. Ma torniamo, Presidente, al metodo del provvedimento: una risposta sbagliata a una domanda sbagliata, dicevo. Chiedersi come fare a evitare o a chiudere e a sanare le procedure di infrazione non è la domanda giusta, secondo me, che sarebbe invece: qual è il veicolo più efficace e utile, quello adatto, il più congeniale per sanare le procedure di infrazione? E qui veniamo alla risposta sbagliata, perché in realtà lo strumento per questo tipo di finalità e per questa esigenza esiste ed è uno dei pochissimi appannaggio della Commissione alla quale appartengo, la affari europei, che, ramo cadetto, maneggia due provvedimenti principalmente: la legge di delegazione e la legge europea. - per il suo tramite, Presidente - della legge europea, lo strumento fatto apposta per questo tipo di finalità, ancora nessuna traccia - forse, si vedrà - depauperando, anzi espropriando la Commissione, dunque il Parlamento, di provvedimenti che fanno la spola e la navetta tra istituzioni europee ed istituzioni italiane e che - ripeto - sarebbero identitari, come usa dire a destra, Mi chiedo: ma se i due provvedimenti cardine del nostro lavoro di commissari vengono meno, che ci stiamo a fare? *(Applausi).* A che serve la Commissione affari europei, che pure nella scorsa legislatura abbiamo difeso con le unghie e con i denti, rivendicando lo specifico europeo in Parlamento? Dite di essere convertiti all'Europa? Fate funzionare la Commissione affari europei, fatela lavorare. Consentiteci di usare gli strumenti a nostra disposizione, dateci la legge europea. Sul merito, Presidente, ieri nel lavoro in Commissione (vado in ordine sparso) abbiamo visto la maggioranza negare maggiori risorse e investimenti ai Vigili del fuoco. Inviterei chiunque di voi, i più scettici sul cambiamento climatico, a uscire da questa bella Aula climatizzata e a farsi un giro per strada, dove vivono le persone e arde l'estate più bollente di sempre. Rivolgo la mia, la nostra solidarietà ai Vigili del fuoco *(Applausi)*, chiamati a lavorare sulle forze in quest'estate rovente. Sappiate che i vostri fondi non sono stati bollinati; nell'Italia dei roghi, la destra scommette sul ponentino, magari funziona. Abbiamo visto la maggioranza votare contro il riconoscimento dei docenti delle scuole paritarie, dopo anni e anni, con la destra che si stracciava le leggendarie vesti sulle paritarie. *(Applausi)*. Ieri in Commissione - come ha ricordato benissimo la senatrice Malpezzi - neanche la terminologia gli andava bene. Per la destra, sappia che, se insegni in una scuola paritaria, sei un docente di serie B, vali di meno: rassegnati. Abbiamo visto la maggioranza trasferire al TAR il diritto di un ricorrente di fronte a un provvedimento di respingimento alla frontiera ad avere un pronunciamento di un giudice ordinario, uno slittamento uno slittamento sul piano dei diritti con conseguenze assai rilevanti, una delle misure più insultanti di questo decreto-legge, l'amministrativizzazione di un diritto e penso alla battaglia che ha fatto per noi Tatiana Rojc sul tema dei visti, con un emendamento che è sparito, diciamo lo abbiamo detto, lo ha detto il senatore Martella a più riprese nella discussione degli emendamenti - il provvedimento è totalmente slegato dal merito, calato all'ultimo minuto in Commissione, figlio di nessuno, tanto che sotto c'è uno scontro tra il ministro Fitto, il plenipotenziario della *premier* che mi spiace non sia presente, e il ministro Urso, uscito scornato da questa decisione del Governo, ma questa ve la vedete Quello che invece impatta sugli italiani è un provvedimento che, non solo il Partito Democratico, ma le istituzioni territoriali di Taranto ritengono un colpo di mano, con pesanti effetti sul tema della decarbonizzazione, il solito accentramento nelle mani del solito ministro Fitto - ma quante ne vuole, Ministro, quante ne vuole? *(Applausi)* - e con una sconfessione di quanto fatto l'altro ieri sotto il Governo Draghi,

e questo provvedimento discrezionale, erratico, rabberciato - se ne farà una ragione il presidente Terzi Di Sant'Agata, che ieri ne difendeva la coerenza e ha tutta la mia solidarietà umana - ne è la fotografia più chiara e senza filtri. Certo la natura di questa destra sta lì, per per la sua storia, per una classe dirigente che mi pare un po' in difficoltà - per usare un eufemismo - nel salto dimensionale e quindi ogni tanto, spesso, anzi, riemerge, si riaffaccia e - come si dice a Roma, dalle mie parti - si ripropone come i peperoni. Non voglio però rimproverarvi una metamorfosi repentina e spregiudicata e non penso certo che alcuni guai con con l'Europa e con il *mainstream* europeo nascano tutto d'un botto con il Governo Meloni: sarei più stupido che ingiusto. Tuttavia, scusatemi, per amore di verità - non è un inciso, ma è il punto sull'Europa - credo, ad esempio, che l'affidamento della responsabilità del PNRR, passato dal MEF al ministro Fitto, sia stato sbagliato, perché in tutta Europa è il Ministero delle finanze a gestire il PNRR *(Applausi)*. Gli affari europei, infatti, non avevano e non hanno ancora il personale, i decreti, le risorse, la forza e l'autorevolezza di andare in Europa come dovrebbe andare un Paese come l'Italia. Lo dico con grande rispetto e considerazione personale per il ministro Fitto - mi dispiace, ministro Ciriani, che non sia presente - sempre capace peraltro di scaricare a terra gli eroici furori dell'opposizione, con una retorica languida, rotonda, che qui funziona e molto, lo ammetto, non so però quanto a Bruxelles. Avere perso tutti questi mesi è stato un danno per il Paese, un'inutile perdita di tempo che si è scaricata e si scaricherà, non solo sulle rate del Piano, ma sulla sua efficacia e sulla sua utilità complessiva. Non sto dicendo che sia una gigantesca unica occasione perduta, tutt'altro; però, se posso, vi abbiamo dato una disponibilità sincera a collaborare in Parlamento e a fare il massimo perché il PNRR sia e possa ancora essere uno straordinario successo. Non si tratta solo di venire ogni tanto in Aula o in Commissione a scambiarci malizie o convenevoli; si tratta di riconoscere che questo Piano è uno sforzo collettivo e un'opportunità straordinaria per il nostro Paese. Posso dire, Ministro, che nella vostra narrazione - oso dire nel vostro impegno - questa spinta, questa urgenza è completamente assente? Posso dire che, nel fastidio verso le critiche, vedo una piccata versione del lasciateci lavorare, che non serve a nessuno, non a noi, non a voi e, soprattutto, non agli italiani? che, se il commissario Hahn vi chiede di correre sull'attuazione, la cabina di regia non è esattamente la risposta giusta? La scommessa comune dovrebbe essere la stessa: presto e bene, presto e bene, se possibile con uno sforzo quotidiano a far comprendere come dietro l'ostico acronimo PNRR si nascondano il parco sotto casa, la fibra per vedere i film, i mezzi per spostarsi in città e fuori, le strade, il rinnovamento delle scuole, gli asili nido *(Applausi)* che liberano il tempo delle persone, ma non lo state facendo, non lo vedo, Ministro: beato lei, se lo vede, noi no. Oggi questa responsabilità è vostra, ve l'hanno consegnata gli italiani, che capiscono bene che perdere tutte queste opere, dilapidarle, sprecarle sarebbe una catastrofe nazionale, un fallimento, non solo italiano, ma europeo. La stanga richiamata dal presidente Mattarella per tutti è esattamente questa, come stanno facendo altri Paesi, valorizzando e andando a vendere in giro per il mondo le trasformazioni rese possibili dal PNRR come occasione di investimento, di conversione, di crescita intelligente. Dovreste e dovremmo avere la fame del Dopoguerra, la lena del boom, la capacità di risalire degli italiani, unica al mondo. Quello che vediamo, Ministro, sono mezze scuse, statistiche per dire che anche gli altri sono nelle peste, vaghe rassicurazioni, disturbo verso le critiche e i richiami, pletoriche riunioni in sala verde, ma non funziona così a Bruxelles. Non funziona così, ma non per un complotto globalista o per colpa degli eurocrati, che anzi mi pare si dispongano ad aiutare e molto, ma per la vostra difficoltà, la vostra lentezza, la vostra reticenza a entrare in gioco, a difendere - come fanno i grandi Paesi - i nostri interessi, quelli dei cittadini, in maniera decisa, concreta, collaborativa e intelligente. Ministro, in Europa abbiamo un gentiluomo che si chiama Paolo Gentiloni. *(Applausi)*. Ho avuto il raro privilegio di collaborare con lui a Palazzo Chigi. Conosco il suo decoro, la sua dignità, il suo senso delle istituzioni e il suo sentimento per l'Italia. Ieri, in un'intervista a un vostro Sottosegretario, uno di quelli (non pochi) che vi fa e ci fa danno, ho letto un suo scomposto attacco al nostro Commissario italiano. Va bene, manca l'ABC, ma se non si distingue tra le persone e le istituzioni che quelle persone rappresentano, tra amici e nemici, non state facendo un buon servizio al vostro Governo, all'Italia e agli italiani. Fidatevi. Potrei stare qui a ricordare i ritardi, la terza rata, la quasi certezza della quarta rata che arriverà nel 2024: non è questo il problema. Quello che dico è che non potete stare a mezza costa, europeisti ma riluttanti, sospesi tra il prima lepenista e le sirene dei popolari europei. Se il vostro cambiamento è autentico, dimostratelo. Avete lo strumento giusto, il PNRR, il MES - mi scuserà il senatore Borghi - e il negoziato sul Patto, la solidarietà Atlantica. Ma, se venite risucchiati dal passato, sarete pietrificati e sarà una catastrofe per tutti. Credere nell'Europa; per essere credibili in Europa bisogna crederci nell'Europa. Signor Presidente, concludo: cominciate a fidarvi del Parlamento e dei suoi strumenti, come la legge europea. Prendete impegni, invece di porre mano alla decretazione d'urgenza, perché la perdita di tempo che questo comporta è un danno che non possiamo permetterci, perché l'orizzonte di un Paese come il nostro è più ampio di così, più largo di così, più alto di così, perché siamo un grande Paese e in Europa contiamo. A nome del Partito Democratico, signor Presidente, per tutto questo, annuncio la nostra astensione sul provvedimento. Per le norme sull'Ilva

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare concerne la conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, che prevede l'adozione di provvedimenti necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012. La finalità del decreto-legge è appunto nella necessità di ridurre al più presto il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e l'urgenza di evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle già esistenti. Ricordo che al momento dell'insediamento del Governo Meloni il numero delle procedure di infrazioni pendenti era di 83, a fronte di una media europea di 73. Da allora ne sono state chiuse ben 11, mentre altre 10 sono state aperte in relazione a risalenti situazioni di non conformità. Alla data odierna, dunque, il numero delle procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati EUR-Infra, è di 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento delle direttive, a fronte di una media europea di 66. Con il decreto-legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che consentiranno di agevolare la chiusura di un rilevante numero (circa 35) di procedure di infrazione, nonché di prevenirne di nuove, consentendo in numerosi casi di evitare di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie a carico del bilancio statale. Si tratta di una quota di adempimenti ben superiore ad analoghi interventi effettuati in passato e tutti fanno seguito a positive interlocuzioni con la Commissione europea, ad ulteriore dimostrazione del costante e proficuo dialogo che il nostro Governo sta portando avanti con successo con le istituzioni europee. Quindi, un ottimo lavoro del Ministero degli affari europei e del ministro Fitto in particolare, il quale anche in questa circostanza ha dimostrato la sua competenza e al quale, anche per la sua costante disponibilità al confronto parlamentare, va il nostro apprezzamento. Entrando nel dettaglio dell'articolato, ricordo che esso si compone di 27 articoli interessanti varie tematiche, con importanti provvedimenti spesso attesi da anni. Vorrei citare l'articolo che reca modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, introducendo un termine entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità della banca di adempiere ai rimborsi dei dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria: si tratta quindi di un'ulteriore tutela dei risparmiatori. Cito poi la norma che prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro i quali abbiano risieduto e svolto la propria attività in Italia: è un esempio di una disposizione che va a sanare una procedura che risale al 2014. Ricordo pure quanto previsto in tema di pubblicità nel delicato settore sanitario, per garantire una comunicazione funzionale e allo stesso tempo che non possa determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari con messaggi a carattere attrattivo e suggestivo. Questo sempre a tutela sempre dell'interesse dei pazienti. poi evidenziare anche le importanti norme di carattere ambientale, a dimostrazione della concreta e mai ideologica attenzione di questa maggioranza per l'ambiente e la salute. In particolare, ricordo gli articoli che recano: l'istituzione dei fondi per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media del radon - il gas nobile prodotto dal decadimento dell'uranio naturale, altamente cancerogeno - superi nell'aria il livello di riferimento; la definizione delle priorità di intervento, come pure la prevenzione e il contenimento del radon negli ambienti chiusi. le misure in materia di circolazione stradale, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, con le modifiche del codice della strada. Le novità introdotte dal Governo riguardo l'Ilva di Taranto consentono di proseguire nell'attività di modernizzazione dello stabilimento siderurgico (a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da qualche opposizione), in attuazione del piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, coniugando la continuità dell'attività produttiva con la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e lavoratori. Anche sulle tematiche del lavoro troviamo importanti novità: l'attesa normativa per il personale a tempo determinato delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con un risultato peraltro condiviso con l'opposizione; il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori, conformando così la legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato per la categoria del personale discontinuo del Corpo. Sempre con riguardo ai Vigili del fuoco, ricordo le disposizioni sull'assetto del personale volontario, con una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di Vigili del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari discontinui. Sul tema della scuola ricordo le importanti e attese disposizioni in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato per tutto il personale delle istituzioni scolastiche; le disposizioni in materia di carta elettronica del docente, con l'estensione del beneficio cui è associato un *bonus* di 500 euro anche ai docenti con contratto di supplenza annuale. Significativi poi i provvedimenti previsti in materia di giustizia e sicurezza: tra questi, l'attuazione del regolamento dell'Unione sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione. ancora le disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti per consentire l'interoperatività dei sistemi informativi europei per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. Di rilievo anche le disposizioni sul settore energetico, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Abbiamo introdotto una norma finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, che consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse, a tutela quindi dell'utenza. Sempre sull'energia, segnalo il riordino della normativa sull'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. menziono la norma a tutela dei produttori agricoli in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola ed alimentare. In conclusione, colleghi, questo importante provvedimento conferma la volontà del Governo di ridurre significativamente il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti sull'Italia avvicinandoci alla media europea di procedure per Stato membro. Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati. È importante sottolineare come ogni disposizione contenuta sia stata concordata preventivamente con la Commissione: un'ulteriore prova di un dialogo costruttivo e costante con le istituzioni europee. Certamente, colleghi, questo provvedimento rappresenta un altro tassello di un complicato lavoro che il nostro Governo sta svolgendo con autorevolezza in Europa. A tal proposito, permettetemi di evidenziare la recente firma del *Memorandum* d'intesa fra l'Unione europea e la Tunisia. un risultato, un successo, fortemente voluto e ottenuto dal nostro Presidente del Consiglio *(Applausi)*, che rappresenta solo una parte di un'ampia strategia di accordi tra Unione europea e Nazioni africane, in cui si coniughi la cooperazione sul contrasto ai trafficanti a una forte accelerazione nei rapporti economici e nelle politiche di approvvigionamento di energia sostenibile. Così pure la recente importante apertura della Commissione al progetto della zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno, in una prospettiva di lavoro e sviluppo del nostro meridione, non più di assistenza improduttiva. colleghi, a dispetto di quanti prevedevano un'Italia esclusa ed emarginata in Europa, con il Governo Meloni l'Italia è protagonista, a testa alta e con le carte in regola *(Applausi)*. È per questi motivi che annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso *weekend* ho fatto visita a un mio concittadino gravemente malato, affetto da lesioni cerebrali causate da un'ischemia e con seri problemi cardiaci. Si chiama Andrea. Ebbene, nonostante le avverse condizioni di salute, nella morsa di un caldo cocente che sta flagellando l'Italia, quest'uomo, sotto sfratto a breve, dovrà abbandonare la propria abitazione, contando solo su una pensione di 300 euro al mese. Si è avvicinato a me e mi ha detto: «Cosa devo fare per sopravvivere? Sono solo e disperato». Mi ha implorato più volte, spiegandomi che ha spesso fatto richiesta di un alloggio popolare, senza ricevere alcuna risposta. Ebbene, la sua storia è solo un tassello di un *puzzle* più grande, che unisce lungo lo stesso solco migliaia di cittadini della mia terra. Basti pensare che, solo negli ultimi mesi, oltre 500 famiglie di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno fatto domanda per ottenere un alloggio di edilizia pubblica popolare, il che accende un riflettore sull'emergenza abitativa che investe l'area vesuviana. A ciò si aggiunge lo stato di pericolo in cui vivono migliaia di residenti, costretti a vivere in case o palazzi fatiscenti, pericolanti e degradati. Purtroppo è notizia di pochi giorni fa che più di 80 persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito di un crollo che ha visto protagonista un edificio di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli: un episodio drammatico, che fortunatamente non ha provocato vittime, ma ha creato un'ulteriore emergenza abitativa. Onorevoli colleghi, l'emergenza abitativa è una realtà che va affrontata con soluzioni rapide e concrete, nel rispetto dei tanti cittadini che versano in condizioni di povertà. di povertà. Per questo motivo sto lavorando ad un disegno di legge che reca proprio l'obiettivo di introdurre nuovi strumenti di sostegno alla rifunzionalizzazione delle aree marginali e alla lotta contro l'emergenza abitativa. Onorevoli colleghi, fare finta che certi problemi non esistano, indossando i paraocchi, non aiuta a risolverli, ma li amplifica. Per questo motivo, già nelle prossime settimane presenterò la mia proposta di legge. Signor Presidente, voglio ricordare anch'io la figura di Andrea Purgatori, il giornalista che purtroppo ci ha lasciati, questa mattina, dopo una breve malattia. Andrea Purgatori è stato un personaggio importante, non soltanto per l'informazione italiana, ma penso per tutti gli italiani. Le sue inchieste e il suo lavoro giornalistico sono stati probabilmente parte della nostra educazione civile, e non soltanto della nostra informazione, toccando spesso questioni che

La sua inchiesta sulla strage di Ustica, per esempio, credo che non soltanto sia stata un esemplare momento di informazione, ma abbia anche costituito un vero e proprio baluardo a difesa della verità e a difesa dei fatti. La voce di Purgatori, la sua capacità di condurci dentro la complessità e dentro anche i misteri di quelle vicende, di quella vicenda in particolare ma non solo, sono servite a dare a tutti noi anche una certa sicurezza rispetto alle scuse e scuse e alle menzogne evidenti che venivano avanzate da più parti. Quindi, credo che il suo sia stato un lavoro fondamentale per la nostra comunità nazionale e per la nostra coscienza civile. Voglio ricordare anche il suo impegno ambientalista. Purgatori è stato anche presidente di Greenpeace. Però, c'è una cosa che vorrei in particolare sottolineare: tutto questo lavoro così intenso, questo lavoro così ficcante, questo lavoro così efficace è sempre stato svolto da Purgatori con un estremo garbo, con un'estrema civiltà, con un modo di porsi rispetto agli ascoltatori estremamente rispettoso. *(Applausi)*. Nel grandissimo rumore, nel grandissimo *can can* che è la nostra televisione, mi permetto di dire che spesso anche i programmi di approfondimento giornalistici fanno a gara per alzare il volume al massimo e per ottenere la massima attenzione sulla forza del rumore e non sulla forza dei fatti; servant*, un servitore del nostro senso di civiltà, che ha portato avanti con la tenacia, con l'approfondimento e con lo studio il suo lavoro e non facendo leva sullo scandalo, sul rumore e sul fracasso, io credo che sia stato un duro colpo per il Paese, perché abbiamo perso non soltanto un grande lavoro di qualità, ma anche una lezione di stile e una lezione di civiltà del dibattito, che mai come in questo momento ci mancherà. Quindi, addio Purgatori, ci mancherai.

Signora Presidente, anche io esprimo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Andrea Purgatori. Oggi il nostro Paese perde una voce libera e coraggiosa; perde un uomo che era tante cose. Andrea Purgatori era un giornalista d'inchiesta, inviato storico del «Corriere della sera», autore di *reportage*, regista, sceneggiatore, scrittore, conduttore di trasmissioni televisive. È stato anche - come ricordava il collega Scalfarotto - presidente di Greenpeace. Andrea si è occupato di tante inchieste su temi scottanti. Si è occupato di mafia, di terrorismo negli anni di piombo, si è occupato del caso Moro, della strage di Ustica. Ha raccontato tante guerre per questa sua capacità, per questo suo coraggio, anche per il rigore nelle sue inchieste, per il rigore con cui cercava la verità, Andrea ha ottenuto tanti premi: il Nastro d'Argento nel 1992 per il film «Il muro di gomma» sulla strage di Ustica, il premio Hemingway di giornalismo nel 1993, il Globo d'Oro nel 1994 e nel 2009, il premio Amidei per il film «Fortapàsc», che parlava di Giancarlo Siani. Oggi Andrea manca alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Andrea mancherà a chi, come me, è cresciuto con quella sua voce calma e rassicurante, che ti guidava verso la verità. Andrea mancherà ai tanti giovani giornalisti che in lui avevano un modello da seguire e ai tanti giovani che con lui hanno condiviso tante battaglie ambientaliste. mancherà soprattutto ai suoi colleghi e al giornalismo di inchiesta, che è sempre fondamentale per la ricerca della verità, indipendentemente dal potente di turno. Anche per lui noi, come forza politica, continueremo a difendere il giornalismo di inchiesta.

ventiquattro anni, la corte d'assise ha condannato due responsabili per l'omicidio di Emanuele Scieri, giovane allievo paracadutista siracusano che fu trovato morto il 16 agosto 1999 e rispetto al quale una vicenda complessa di silenzi e di reticenze che è durata anni e che è passata per diverse archiviazioni è stata poi illuminata da una Commissione parlamentare fortemente voluta dal Partito Democratico, ma estesa poi a tutte le altre forze politiche, che con fatica, con 45 audizioni e il lavoro instancabile della sua Presidente, l'onorevole Sofia Amodio, ha portato ad una mole di evidenze tecniche che oggi, per riconoscimento esplicito del procuratore che se n'è occupato, hanno permesso di conseguire una prima condanna. In quella circostanza - mi piace ricordarlo anche oggi, per una triste coincidenza

In quel caso, riguardava il nonnismo e la violenza nel mondo militare e uno degli aspetti tragici che poi quella Commissione d'inchiesta rivelò fu la circostanza che probabilmente

che era stata indotta appunto da alcune azioni violente di nonnismo, permettevano di salvare quella vita, visto che la morte probabilmente è sopravvenuta, com'è stato riconosciuto, dopo diverse ore.

di gomma - ma anche l'idea che uno Stato e una Patria sono forti anche quando rivelano le proprie fragilità e anche quando hanno il coraggio di dimostrare una verità scomoda; anzi, lì forse sono più Stato e più Patria che altrove. Mi preme allora ricordare qui che in quella pressoché unanime decisione della commissione di giustizia, ci fu solo un'astensione giustificata dalla motivazione, secondo la dichiarazione del portavoce, che in quel caso si trattasse in realtà di un pregiudizio della sinistra nei confronti della brigata Folgore. Queste furono le parole dell'allora portavoce di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, che mi dispiace non sia qui presente, che non votò e si astenne dalle conclusioni di quella commissione che invece oggi ha portato ad una prima verità giudiziaria. Quello che ci resta e che va ricordato a quest'Assemblea è che quando queste persone muoiono

la Patria anche riportando in vita la dignità delle persone che ne sono vittime, in questo caso Emanuele Scieri, figlio amato, siracusano, mai dimenticato, giovane allievo paracadutista, ragazzo italiano, patriota.

ricerca (MIUR), tramite la ministra, collega Bernini, ha fatto slittare una graduatoria su messa a norma della scuola e ci viene finanziata con fondi PNRR una riqualificazione di oltre 500.000 euro. Ottima notizia, se non fosse che abbiamo circa settanta giorni per progettare, bandire gara e assegnare. È una follia, siamo a fine luglio. Nel frattempo, va considerato che è cambiato il codice degli appalti e la nostra centrale unica di committenza non farà gare fino alla fine di settembre.

Sarebbe bastata una proroga e avremmo potuto sistemare la scuola. L'intervento precedente del senatore Sensi faceva proprio riferimento a questo. Il PNRR dà a questo. Il PNRR dà finanziamenti che servono proprio per le persone, per le scuole, per la carne viva delle persone. Disporre uno slittamento di queste liste e non dare poi il tempo fisico per progettare e bandire le gare è veramente una follia che noi parlamentari non possiamo permetterci e dovremmo fare in modo che il Governo possa dare una proroga affinché i fondi del PNR vadano in porto come si deve.